L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

790.000 incidenti e 1.050 decessi. Bisogna invertire il *trend* e per farlo è necessario provvedere a sanare le tante criticità che ancora si registrano

Un punto di partenza è certamente il decreto legislativo n. 81 del 2008 il cosiddetto Testo unico sulla sicurezza - che, con le successive modifiche ed integrazioni - mi riferisco, prima di tutto, al decreto legislativo correttivo n. 106 del 3 agosto 2009, le cui norme sono entrate in vigore il 20 agosto successivo ha definito un *corpus* organico per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma se il Governo non provvederà, ci auguriamo in tempi brevi, ad emanare i decreti attuativi, molte disposizioni che disciplinano gli aspetti di dettaglio resteranno sulla carta. La gran parte dei decreti, infatti, non è ancora operativa. Dagli ultimi dati forniti dal Ministero del lavoro risulta che nella seconda metà del mese di gennaio è stata programmata la discussione su alcuni commi dell'articolo 6 del Testo unico, relativo alla Commissione consultiva permanente per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per procedere in particolare alla rielaborazione della procedura standardizzata per la valutazione dei rischi, per la qualificazione delle imprese, per i modelli di gestione della sicurezza, per la formazione in materia di salute e sicurezza. Su aspetti fondamentali, dunque, i provvedimenti normativi non sono ancora stati definiti. Nell'effettuare, a nome del Gruppo del Partito Democratico, la dichiarazione di voto sulla seconda relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione d'inchiesta, colgo l'occasione per ribadire, soprattutto sulla base di quanto è emerso nel corso dell'indagine e delle audizioni della Commissione, che deve venire principalmente dal Governo la spinta ad assicurare l'attuazione della riforma prevista dal Testo unico sulla sicurezza.

in modo da offrire a tutti i soggetti preposti alla tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - dalle imprese ai lavoratori agli enti istituzionali - anche una applicazione uniforme delle disposizioni. il Governo deve impegnarsi a potenziare e promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, attraverso campagne di informazione mirate, ma soprattutto attraverso un'adeguata formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Ministro dell'istruzione e quello del lavoro, accogliendo una proposta avanzata dal Partito Democratico, ma condivisa anche da altre forze politiche, si sono detti favorevoli ad inserire l'insegnamento sulla tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dei programmi della scuola dell'obbligo e dell'università. Ecco, riteniamo che si debba tener fede a questo impegno, garantendo risorse adeguate, indirizzi omogenei e insegnanti qualificati. Allo stesso modo, è opportuno introdurre forme di incentivazione per premiare le imprese virtuose che investono sulla sicurezza dei propri dipendenti, attraverso sgravi ed ed agevolazioni fiscali e contributive, nonché proseguendo con la concessione di incentivi per rottamare e mettere in sicurezza macchine, attrezzature, impalcature, ponteggi e piani di lavoro, spesso obsoleti, la cui efficienza è essenziale per prevenire infortuni che spesso, purtroppo, si rivelano mortali. Un altro fronte sul quale si registrano ancora criticità è quello relativo agli appalti. Occorrono iniziative legislative ed amministrative, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e della libertà di impresa, per intervenire sui ribassi d'asta. Bisogna porre limiti precisi: il ricorso al massimo ribasso d'asta, come da noi segnalato in un apposito ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato il 21 ottobre dello scorso della relazione annuale, non può continuare a costituire uno dei principali criteri di valutazione delle offerte, dal momento che esso rappresenta un canale privilegiato di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia del Paese. Si può cominciare a porre argine al dilagare di quello che appare un vero e proprio cancro da estirpare, soprattutto in alcune zone del Paese, come il Mezzogiorno, accrescendo la qualificazione delle imprese e contenendo la pratica dei subappalti. L'obiettivo è quello di estendere quanto più possibile, anche al settore privato, le garanzie e i controlli vigenti nel settore pubblico. A proposito di misure di incentivazione alla sicurezza sui cantieri edili, la Commissione ha valutato una serie di proposte, a partire da specifici incentivi per sostenere le imprese che agiscono in modo virtuoso su questo fronte: il premio di sicurezza, ad esempio, da corrispondere previe specifiche verifiche del responsabile del procedimento alle ditte aggiudicatarie degli appalti che abbiano applicato tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in tema Ancora, nel caso in cui dagli accertamenti risulti che le imprese abbiano adottato nel proprio sistema organizzativo adeguate politiche di tutela dell'incolumità e della salute dei propri lavoratori - a partire dalla formazione,

sempre ai fini di incentivare la cultura della sicurezza attraverso un miglioramento continuo delle condizioni dei luoghi di lavoro, istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo per la sicurezza e la salute dei lavoratori denominato Fondo per la vita.

Per quanto ci riguarda - e concludo - riteniamo necessario che il miglioramento delle condizioni di sicurezza nel cantiere in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto degli appalti debba essere inserito tra i criteri di valutazione delle offerte presentate per aggiudicarsi l'appalto della gara. Il punteggio da assegnare a tale criterio non potrà essere inferiore a quello, considerato tra i più importanti ai fini dell'aggiudicazione delle gare, dei tempi di esecuzione dei lavori. Si tratta di proposte che mirano al conseguimento dello stesso obiettivo, ma sono animate anche dal medesimo principio ispiratore, che è quello di una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle imprese, rispetto alla necessità di procedere con atti concreti al potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro. In tal modo, in un'ottica di sempre più stretta collaborazione (a ciò invitati di continuo anche dal Presidente della Repubblica) tra tra istituzioni ed imprese, si riuscirà a sbarrare il passo alla criminalità organizzata - purtroppo spesso presente, attraverso ditte collegate o espressione diretta dei *clan* - che vince presentando offerte solo apparentemente vantaggiose, per poi lucrare sulla pelle dei lavoratori. pratiche inaccettabili in un Paese che voglia dirsi civile, il quale non può tollerare oltre le continue morti sui cantieri e sui luoghi di lavoro. Il Paese attende un'azione che rappresenti

sento il dovere di porgere un ringraziamento sostanziale allo stesso presidente Tofani. Lo faccio non solo a nome del PdL, ma di tutti i membri della Commissione, con i quali abbiamo lavorato in sinergia, pur mantenendo visioni distinte su specifiche problematiche. Il nostro fine è stato quello di perseguire la meta comune, di arrivare ad "incidenti zero", e quindi ad un numero Ringrazio inoltre il ministro Sacconi, sempre disponibile ad ogni audizione ad informare ed illustrare il programma e le azioni del Governo sulla materia di contrasto e prevenzione, nonché sulle risorse impegnate o da impegnare. Condividiamo l'azione del Governo, esplicitata nell'intervento del Ministro, che sta lavorando alla attivazione del Testo unico, superando anche quelle lentezze dovute ai numerosi adempimenti, comprese le concertazioni previste nel decreto medesimo. Ci auguriamo che il Governo velocizzi l'emanazione e solleciti fattivamente le Regioni nell'azione di controllo, contrasto, formazione ed informazione che loro compete. L'unanimità raggiunta sulla relazione posta oggi al vaglio di quest'Aula, così come la maggior parte dei concetti contenuti nelle tre risoluzioni, indica che un comune sentire sta maturando tra soggetti che, come abbiamo detto, mantengono alcune visioni distinte su specifiche problematiche.

L'unanimità raggiunta sulla relazione posta oggi al vaglio di quest'Aula, così come la maggior parte dei concetti contenuti nelle tre risoluzioni, indica che un comune sentire sta maturando tra soggetti che, come abbiamo detto, mantengono alcune visioni distinte su specifiche problematiche. Rileviamo con soddisfazione che un buon tratto di strada è stato fatto con il decreto legislativo n. 81 del 2008 e con il successivo decreto n. 106 del 2009, rappresentano una tappa importante nella legislazione nazionale. Al controllo, alla repressione e a quella parte di sanzioni inevitabili, oggi si sono aggiunti la formazione, l'informazione e l'incentivo per i virtuosi. Questa rivoluzione culturale...

Vorremmo poi puntualizzare la questione degli infortuni *in itinere*. Se ai 283 casi di morte avvenuti a seguito di infortuni *in itinere* si aggiungono i 303 registrati tra chi lavora per strada, si scopre che dei 1.050 caduti sul lavoro oltre il 55 per cento è imputabile alla circolazione stradale. Questa è una strage nella strage! Inoltre, si ritiene che sia indispensabile ed urgente intervenire anche nel campo degli infortuni domestici, sui quali ha ampiamente relazionato la collega Colli, così come è

l'attivazione del registro di raccolta dati Malprof, che deve essere adottato da tutte le Regioni e da collegare con il SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), che ha lo scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Passiamo ora alla questione degli con la proposta del Governo di assumere adeguate iniziative per la sicurezza del lavoro nel settore degli appalti e dei subappalti, un argomento ampiamente affrontato in Commissione, anche se è chiaro che la prassi degli appalti pubblici al massimo ribasso non risulta di per sé causa di incidenti.

incongruo per rientrare nei costi. Di fronte a ribassi anomali, occorre chiedere la congruità dei prezzi con evidenziati i costi della sicurezza e l'utile d'impresa. Gli istituti preposti controllino che il costo della sicurezza non venga intaccato, sia in riferimento agli appalti che ai subappalti, soprattutto se

Il raggiungimento dello scopo che tutti ci prefiggiamo, cioè la mortalità zero, passa per il coinvolgimento di tutti gli attori e con la collaborazione delle imprese. È la collaborazione la strada che apre le maggiori possibilità perché diminuiscano ancora gli incidenti sul lavoro! Con questo medesimo, convinto, paradigma culturale, sarebbe auspicabile che oggi una convergenza delle tre risoluzioni, come hanno indicato il presidente Tofani ed il ministro Sacconi, L'unità di fondo che ha caratterizzato i lavori della Commissione non cancella sensibilità diverse, ma sarebbe un segnale positivo per tutti se quel comune sentire prendesse oggi corpo con un atto condiviso. Siamo convinti che la sfida di civiltà per la sicurezza del lavoro sarà vinta davvero solo quando verrà completato quel ribaltamento di mentalità che abbiamo intrapreso, così che nessuno dovrà più mettere in pericolo la propria vita per guadagnarsi il pane.

Bugnano ed altri, il parere è contrario per quanto riguarda le premesse e il considerato

alla mozione n. 3, della senatrice Bugnano ed altri, il parere è contrario per quanto riguarda le premesse e il considerato

Il Governo esprime un parere sostanzialmente conforme a quello del relatore con due osservazioni. relativa alla motivazione della non condivisione delle considerazioni preliminari che sono nelle seconda e nella terza proposta esse rinnovano una critica che più volte l'opposizione ha avuto modo di manifestare sull'apparato sanzionatorio, così come corretto dal decreto decreto legislativo prodotto nel corso di questa legislatura, ed evidentemente il Governo non può accogliere questa considerazione. Per quanto concerne invece contenuti nei dispositivi delle due proposte di risoluzione, il Governo si rimette al relatore e all'Aula con un'unica avvertenza: ricorrono alcuni oneri di finanza pubblica che possono essere essere soddisfatti solo compatibilmente con l'andamento generale dell'economia e del bilancio dello Stato.

Ha facoltà

Ha facoltà di parlare il senatore Tonini per illustrare la mozione n. 359. Signora Presidente, insieme al collega Ceruti e a quasi tutti i colleghi del Gruppo del Partito Democratico abbiamo presentato nei giorni scorsi la mozione n. 359 sulla persecuzione dei cristiani, a partire naturalmente dall'allarmante intensificarsi di episodi di assoluta gravità

per il solo fatto dell'appartenenza a una religione. Questo fenomeno sta diventando allarmante nel suo ripetersi e nel suo intensificarsi ed ha provocato da parte nostra la richiesta di un'attenzione specifica da parte dell'Aula del Senato, come peraltro in via parallela è stato fatto anche nell'altro ramo del Parlamento con un'analoga iniziativa Queste violazioni sistematiche e ripetute della libertà religiosa sono allarmanti, non solo per i credenti, ma, ritengo, per tutte le persone che hanno a cuore la dignità dell'uomo ed i valori di libertà e di rispetto dei diritti umani fondamentali, anche perché la libertà religiosa è storicamente la madre di tutte le libertà. Ricordo che in Europa i principi fondamentali di libertà nacquero anche nel tentativo di uscire dalla lunga, buia stagione delle guerre di religione europee europee e che gli Stati Uniti d'America sono nati anche ad opera di quei Padri Pellegrini che, fuggiti dall'Europa perché perseguitati sul piano religioso, fondarono il primo degli Stati americani sulla base del principio della libertà religiosa. Quindi, il principio della libertà religiosa è un principio fondante per tutti i diritti umani e per tutte le confessioni religiose.

hanno un preciso obiettivo che deve essere compreso e cioè vogliono utilizzare la religione come combustibile per una guerra fondata sull'ideologia dello scontro di civiltà e sulla contrapposizione tra comunità in base alla loro appartenenza religiosa. Questo disegno deve essere condannato in maniera ferma da tutta la comunità internazionale e deve essere respinto con la massima determinazione e la massima energia, e la massima energia, evitando di commettere due errori. Il primo è quello di identificare gli attacchi contro i cristiani come espressione della comunità islamica nel suo insieme, quando invece spesso gli attacchi ai cristiani sono il tentativo di componenti minoritarie, fanatiche, fondamentaliste di tipo islamista di accreditarsi come gli unici difensori del vero Islam che per dimostrare questo danno vita ad atti di aggressione nei confronti delle comunità cristiane.

Noi sappiamo che c'è un Islam che cerca la sua strada di ingresso nella modernità e di dialogo con l'Occidente, che crede fortemente nella società multireligiosa, nella tolleranza e nella convivenza tra le comunità religiose. L'Egitto, da questo punto di vista, è una delle Nazioni che più hanno dato esempio positivo nel passato

da 2.000 anni, come avamposti della società occidentale. I copti egiziani sono più egiziani di tutti gli egiziani: non sono qualcosa di estraneo,

i cristiani, anche i cristiani perseguitati, come una sorta di avamposto occidentale in Paesi antioccidentali! Non è così.

sulle orme di Giovanni Paolo II, che scelse questa modalità di testimonianza proprio per scongiurare il pericolo che le tensioni, in particolare in Medio Oriente, potessero trasformarsi nell'innesco di uno scontro di civiltà e di una guerra di religione. La religione è uno dei segni del secolo nel quale siamo entrati - resta un elemento fondamentale dell'esistenza umana e della convivenza umana e civile. Tutte le teorie che immaginavano un superamento della religione come se quest'ultima facesse parte, in quanto tale, di uno stadio infantile dell'esistenza umana si sono rivelate fallaci. La religione è una dimensione costitutiva dell'essere umano e anche della socialità umana, quindi fa parte della dimensione pubblica oltre che di quella privata dell'essere umano. Proprio questa sua forza è una grande responsabilità per la religione, perché naturalmente la religione, essendo questa grande energia e questo grande elemento di forza all'interno delle comunità umane, può essere un potentissimo fattore di convivenza, ma può anche essere un potentissimo fattore di scontro, di violenza, di intolleranza. Quindi credo sia quanto mai utile ed opportuna, da guardare con grande attenzione e con grande interesse, la proposta di papa Benedetto XVI di dar vita a questo incontro tra le religioni per la pace. la pace. Credo che analogamente, nella comunità internazionale, nel suo versante civile e politico, si debba fare ogni sforzo perché l'attenzione ai temi della tolleranza, della convivenza religiosa e della libertà religiosa come diritto fondamentale dell'uomo sia al centro dell'iniziativa politica. Questo chiediamo al Governo con la nostra mozione: gli chiediamo di farsi carico, sia nelle relazioni bilaterali, sia sul piano multilaterale, a cominciare dalla sede europea e dalla sede dell'ONU, di un'iniziativa forte a sostegno della libertà religiosa e contro ogni forma di persecuzione, a cominciare da quelle

la cristianofobia non nasce oggi e nemmeno negli ultimi anni. Siamo qui oggi ad assumere una posizione auspicabilmente forte in quest'Aula parlamentare mossi dall'orrore e dallo sdegno per la strage di capodanno che ha insanguinato Alessandria e per i fatti che sono seguiti, ma sappiamo bene che il fenomeno - con i suoi drammatici risvolti, più o meno noti, troppo spesso dimenticati - affonda in un periodo ben più lungo, non nasce certo in Egitto e - quel che vorremmo chiarire - soprattutto non nasce nelle sue istituzioni. I dati riportati nella mozione presentata dal Popolo della Libertà sono eloquenti: secondo le statistiche dell'OSCE, cento delle persecuzioni religiose nel mondo riguarda i cristiani. E scandagliando la storia delle comunità cristiane nel mondo, nessuno potrà dimenticare, ad esempio, gli "anni di sangue" che si sono inaugurati in Algeria all'inizio dell'ultimo decennio del secolo scorso, i più antichi stermini in Sudan e i più recenti massacri in Nigeria, finanche in queste ore. Potremmo parlare a lungo dell'Iraq o del Pakistan, dell'India o della situazione dell'Iran. Potremmo anche analizzare le tante dimensioni della cristianofobia, che in alcuni Paesi si nutre della copertura e addirittura della connivenza dei rispettivi Governi, mentre in altri - come in Egitto - ha fra le sue vittime i Governi stessi e i loro sforzi di percorrere strade di pace che non confondano mai la religione con la sua terroristica strumentalizzazione. Dunque, signora Presidente, la cristianofobia non nasce oggi; ha invece preso vigore per ragioni geopolitiche quando la fine della Guerra fredda ha modificato gli equilibri del mondo e ha spostato gli assi della conflittualità, accentuando e accelerando la radicalizzazione dell'Islam. ha preso vigore anche per ragioni culturali ed in ciò forse siamo stati complici. Troppo a lungo, infatti, il "politicamente corretto" ha imposto una considerazione ugualitaria di tutte le religioni e soprattutto del loro portato pubblico e ha impedito di affermare che il contributo delle diverse religioni all'affermazione dei diritti umani, della dignità della persona e della sua intima libertà è differente. Troppo a lungo l'Occidente ha consentito che si radicasse quell'"odio di sé" che Benedetto XVI ha definito "strano" e "patologico" perché nell'«aprirsi pieno di comprensione a valori esterni» «non ama più sé stesso» e ha inteso l'incoraggiamento della «multiculturalità» come «abbandono e rinnegamento di ciò che è proprio». Di qui nasce il richiamo della nostra mozione

al principio di reciprocità. Signora Presidente, colleghi, non è difficile rintracciare nella quotidianità dei nostri tempi esempi concreti che rendano le parole di Benedetto XVI molto più che astratti richiami. Quante volte offese al Cristianesimo, ai suoi simboli e alle sue tradizioni vengono tollerate, quando non addirittura applaudite, in nome di una malintesa idea di laicità? Quante volte, per una altrettanto malintesa concezione di accoglienza e non interferenza, si tollerano nei confini della moderna Europa, dell'evoluta Europa comportamenti che calpestano le più elementari dignità della persona, delle donne in particolare, i suoi diritti e le sue libertà? Signora Presidente, stigmatizzando questo doppio metro di giudizio non intendiamo certo proporre una classifica tra le diverse religioni, tutte in quanto fedi degne dello stesso rispetto; tanto meno intendiamo iscriverci o iscrivere il Cristianesimo a una sorta di gara di martirio, o partecipare a una specie di competizione fra vittime. Né crediamo che una forte presa di posizione a difesa dei cristiani nel mondo sia in contraddizione con il sostegno e la promozione della libertà religiosa a tutela delle minoranze in ogni parte del pianeta; al contrario, riteniamo che le due esigenze vadano di pari passo. Con l'odierno dibattito, però, e con la proposta di questa mozione, vorremmo stimolare una riflessione autocritica su un fenomeno che Renè Guitton ha ben spiegato nel suo libro «Cristianofobia», e che determina in Occidente una irricevibile resistenza culturale a riconoscere ai cristiani lo *status* di perseguitati anche laddove il loro sangue bagna la terra. Quasi che i cristiani venissero colpiti non in quanto tali ma in quanto emanazione dell'Occidente. Quasi che, essendo i cristiani in maggioranza in Occidente, non possano essere riconosciuti come minoranza in altre latitudini. racconto del suo viaggio nei luoghi e nei tempi della cristianofobia, Guitton scrive (cito): «Ho capito quanto sia difficile perorare la causa dei cristiani che soffrono nel mondo e quanto essere cristiano, agli occhi di molti, rappresenti un'intollerabile mancanza di buon gusto, per non dire un *handicap* che sarebbe meglio tentare di nascondere». È bene che di questo noi prendiamo coscienza per contrastare l'incendio che divampa, con le armi della consapevolezza e della razionalità. Consapevolezza di noi stessi e razionalità come dato qualificante e universale della natura umana. Ed è ancora una volta il Papa a spiegarci come il non agire secondo ragione sia contrario alla natura divina, e come una ragione sorda di fronte al divino sia incapace di inserirsi nel dialogo vero tra le culture. E se la ragione non può respingere il divino, allo stesso modo l'adesione a una religione - a qualunque religione - non può essere non può essere irrazionale, perché se l'uomo abdica alla propria razionalità arriva a giustificare in nome del cosiddetto indifferentismo e di un malinteso concetto di tolleranza la lesione di libertà e diritti che, come abbiamo visto, può sfociare nella perpetrazione di autentici crimini. È appena il caso di ricordare che dopo quella lezione del Papa a Ratisbona, suor Leonella fu assassinata a Mogadiscio. E che da parte di talune "*élite* illuminate" dell'Occidente non si esitò ad additare per quel martirio, neanche troppo velatamente, non chi lo aveva perpetrato, ma quel Pontefice che - lo ricorda la nostra mozione - aveva messo in guardia contro un terrorismo che strumentalizza l'uomo e anche lo stesso Dio, degradandolo a idolo di cui servirsi. Signora Presidente, colleghi senatori, cade quest'anno il decimo anniversario dell'11 settembre. Dieci anni dopo, dobbiamo constatare come alcune affermazioni che pronunciate allora avrebbero fatto scandalo - basti pensare al pugno nello stomaco inferto da Oriana Fallaci a un assopito Occidente - sono ormai entrate a far parte del senso comune. Ciò è avvenuto da una parte perché certe consapevolezze sono sedimentate, dall'altra perché gli avvenimenti che si sono susseguiti in questo decennio sono di una portata tale che nessuno può più far finta di non vedere. Non si tratta, colleghi, di fare a gara per stabilire chi abbia avuto ragione per primo. Si tratta, alla luce delle nuove consapevolezze imposte dai nuovi drammi della storia, di agire tutti insieme per invertire la rotta.

*(IdV)*. Signora Presidente, cari colleghi, è di ieri la notizia di un nuovo attacco perpetrato in Egitto contro civili cristiani che porta il triste bollettino di un morto e del ferimento di altri cinque in una sparatoria su un treno in viaggio tra Al Minya, nell'alto Egitto, e Il Cairo. Questa tragedia va ad aggiungersi al dramma della morte di 21 cristiani nella notte di Capodanno nella chiesa dei Santi di Alessandria d'Egitto. 22 morti in soli dieci giorni, dunque, ma i numeri sono molto più ampi. Sulla base delle stime dell'ONU sarebbero circa 200 milioni i cristiani nel mondo vittime di persecuzioni e violenze. In tantissimi Paesi mediorientali, arabo-musulmani, tra i quali da ultimo l'Egitto, gli attacchi contro gli edifici di culto cristiani, i fedeli e le loro abitazioni private si stanno purtroppo drammaticamente moltiplicando. Si tratta a tutti gli effetti di un moderno genocidio che la comunità internazionale non solo non può ignorare ma che deve combattere con ogni strumento a sua disposizione. Per questo, come Italia dei Valori, abbiamo presentato questa mozione per chiedere che anche l'Italia, più più di quanto ha fatto sino ad ora, metta in atto «ogni utile iniziativa diplomatica al fine di contrastare con efficacia i soprusi perpetrati, in ogni angolo del mondo, a danno di uomini e donne di ogni razza o etnia, a causa della professione del loro credo religioso». Cari colleghi, è imprescindibile riconoscere che spesso le violenze verso le comunità religiose che costituiscono la minoranza nei Paesi ospitanti sono mosse da considerazioni che non hanno a che fare con i cieli e con Dio ma sono mosse da intenzioni molto più terrene di calcolo geopolitico, di mantenimento o accrescimento del potere militare e culturale da parte dei Governi o dei gruppi organizzati. La storia, anche la più remota, ci ha insegnato come da sempre la religione sia stata utilizzata, strumentalizzata e distorta a fini tutt'altro che ecumenici. Dio e Cesare sono stati spesso sovrapposti in uno stravolgimento del precetto evangelico. Le comunità cristiane locali danno fastidio in Paesi a democrazia ridotta, perché con la loro stessa esistenza diffondono una religione, una cultura e un sistema di vita fondati sul valore assoluto della persona umana, e quindi sulla libertà, sull'eguaglianza di tutti di fronte allo Stato - con gli stessi diritti per l'uomo e la donna - sulla democrazia e sulla giustizia sociale. Ecco perché oggi dobbiamo affrontare la persecuzione dei cristiani con riflessioni e strumenti politici, economici e culturali, senza farci intrappolare in contrapposizioni religiose. Ecco perché nella promozione della «pacifica convivenza tra le diverse comunità religiose nel segno del dialogo del rispetto reciproco», devono guidarci più la nostra Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che il Vangelo e la Bibbia. Dobbiamo riconoscere, cioè, come le violenze siano determinate dalla volontà di «tenere le comunità cristiane in una condizione di isolamento e di estraneità rispetto alle dinamiche sociali, politiche e culturali dei Paesi in cui insistono», oltre che «di impoverire gli Stati, mantenendo la popolazione in situazione di disagio». Nel nostro Paese l'articolo 19 della Costituzione riconosce in modo ampio la libertà di religione, intesa come libertà di fede religiosa e di diritto di ogni individuo di professare la propria fede e di fare propaganda, come libertà di qualsivoglia pratica religiosa, sancendo il divieto di discriminazione tra gli individui a causa della religione professata, garantendo anche la libertà di non professare alcuna fede. La comunità internazionale e l'Unione europea, di fronte a questi continui e ormai sistematici attacchi ai diritti inviolabili degli individui ed in attuazione dei principi ispiratori delle medesime istituzioni, devono necessariamente prendere ed adoperarsi per garantire diritti pari a quelli sanciti dalla nostra Carta, e lo devono fare con strumenti economici, aiutando, con la cooperazione allo sviluppo e con il sostegno finanziario, i Paesi in via di sviluppo, per permettere alla popolazione di uscire dall'indigenza e quindi dalle tensioni interne, per evitare che i cittadini debbano rivolgersi ad organizzazioni fanatiche e violente, che si sostituiscono ai Governi incapaci finanziariamente di fornire servizi sociali, istruzione e sanità, di cui la popolazione ha bisogno, che è la ragione che ha portato al dilagare delle organizzazioni estremiste in Medio Oriente. L'Italia e l'Unione europea devono quindi attivarsi anche con strumenti politici, sostenendo quei partiti moderati che professano la libertà e la pacifica convivenza contro i fondamentalismi; devono inoltre attivare missioni di pace, laddove si intuiscono i sintomi di conflitti latenti. Così come è stato fatto con la partecipazione alla missione internazionale a Timor Est, l'impegno del nostro Paese nelle aree di crisi in ogni parte del mondo è sempre stato sino ad oggi puntuale e concreto, al fine di evitare l'acuirsi di finzioni tra comunità che professano credi religiosi differenti, oltre che per prevenire nuovi motivi di tensione. In questo senso, cari colleghi, dobbiamo continuare con ancora maggiore sforzo. Non è un caso, infatti, che i due più gravi movimenti caratterizzati per la persecuzione e la violenza verso le comunità religiose - il Nazismo e il Fascismo - siano nati proprio quando l'Europa era in ginocchio dopo la crisi economica del 1929. Il germe della persecuzione religiosa è economico, politico e sociale. Ma chiedere il buon esempio agli altri Paesi non basta; l'Italia deve per prima dimostrare tolleranza e accoglienza, lo dico senza alcuna polemica, ma con un vero spirito costruttivo - come stiamo dimostrando di avere oggi - a tutti i colleghi, anche agli amici della Lega,

della nostra capitale e questa ideologia «di rigetto» - se vogliamo anche poco cristiana - non aiutano certo il clima di dialogo e di tolleranza. Servono azioni diplomatiche, dunque, politiche ed economiche forti. Il nostro Governo deve cessare ogni rapporto con i dittatori con i dittatori ed attivarsi immediatamente presso l'Unione europea e l'ONU per riportare la pace e la libertà di culto. Per questo motivo, con la nostra mozione abbiamo chiesto, tra le altre cose, che il Governo promuova presso gli organismi internazionali e sovranazionali a cui l'Italia appartiene efficaci azioni diplomatiche volte all'aiuto degli individui e delle comunità che subiscono violenze legate a motivazioni di ordine confessionale, contribuendo al progressivo sradicamento degli ostacoli alla pacifica convivenza fra i popoli; che esiga un fattivo ed efficace impegno dell'Unione europea affinché assuma una posizione intransigente e definita contro tutte le violazioni del diritto di professare liberamente la fede religiosa e che agevoli le procedure di riconoscimento dello *status* di rifugiato per tutti gli stranieri presenti sul territorio italiano. Voglio chiudere il mio intervento ricordando anch'io il discorso pronunciato da Papa Benedetto XVI, dopo l'attacco ai cristiani ad Alessandria d'Egitto, perché le sue parole riflettono non soltanto i valori di cristiani ma anche quelli laici su cui è fondato il nostro Stato di diritto: «L'essere umano è uno solo e l'umanità è una sola. Ciò che in qualsiasi luogo viene fatto contro l'uomo alla fine ferisce tutti».

Rifiutate anche voi quello che ci accade! Mentre il mondo festeggia l'ultimo giorno dell'anno un terrorista islamico attacca la Chiesa dei Santi in Alessandria d'Egitto; 23 morti e più di 80 feriti. Queste povere persone stavano uscendo dalla messa dopo aver iniziato un nuovo anno con Gesù e nel cuore tanta felicità e speranza per un mondo migliore. Non è il primo attacco che noi cristiani che noi cristiani ortodossi subiamo dai terroristi islamici: nel 2000 bruciarono una intera città prevalentemente cristiana, 21 persone morirono carbonizzate; nel 2010, la notte di Natale, i terroristi spararono addosso ad una comunità che usciva dalla chiesa, sei ragazzi giovanissimi morirono fucilati; ed infine nelle prime ore del 2011 questo terribile fatto. Noi oggi stiamo qui a manifestare per far sentire la nostra voce a tutto il mondo e chiedervi di aiutarci ad ottenere i nostri diritti e a poter professare la nostra religione cristiana in pace».

sulla non grande saggezza di tenere dibattiti identici nei due rami del Parlamento nella stessa giornata, magari per adottare una identica risoluzione. Si ha di fronte una forma di bicameralismo perfetto che talvolta manifesta la propria imperfezione. di un dibattito molto importante ed è bene che i senatori si pronuncino su una materia che riguarda non i cristiani o i credenti nelle religioni del nostro tempo, della storia, bensì le nostre libertà. C'è troppa ipocrisia e troppa leggerezza in merito alla persecuzione dei cristiani nel mondo. Per un certo periodo di tempo si è immaginato si trattasse di reazioni ad atteggiamenti aggressivi, di situazioni di situazioni legate ad antiche e radicate contrapposizioni locali, ma purtroppo non è così. Noi abbiamo a che fare oggi, Presidente, con una intolleranza religiosa che si associa, da una parte, ad un fondamentalismo aggressivo e, dall'altra, ad un atteggiamento e a subculture che inaccettabilmente immaginano di fronteggiare questi fenomeni con relativismo e indifferenza. Le mozioni che sono state presentate sottolineano variamente la debolezza della politica dell'Unione europea, addirittura afona rispetto a fenomeni di questa straordinaria gravità,

parlamentari, si ricorda che la laicità della Repubblica si esprime anche e specialmente nella tutela della libertà religiosa, un valore essenziale nella vita di tutti cittadini. Uno Stato che tacesse di fronte alla violazione di un diritto inviolabile se ne renderebbe immediatamente complice e perderebbe credibilità e autorevolezza. In realtà è un processo politico quello di fronte al quale ci troviamo. Nel Medio Oriente e in aree del vicino Oriente ci troviamo di fronte a tentativi di vero e proprio sradicamento della presenza dei cristiani. In Iraq si è registrata la fuga, determinata da persecuzioni e da paura, di centinaia di migliaia di cristiani che lì hanno vissuto per secoli e per millenni. Credo che su questo non saremo tutti d'accordo in quest'Aula, quindi la mia è una riflessione a titolo personale, ma non c'è dubbio che oggi dobbiamo fare una riflessione amara sugli sviluppi della guerra in Iraq per quanto riguarda la coabitazione tra religioni. Posso testimoniare qui pubblicamente quello che ho ascoltato in quegli anni,

di diventare anche una catastrofe religiosa». Quel santo aveva chiara la percezione della minaccia che una convivenza delicata e difficile, di quell'evento, potesse saltare definitivamente. Molti di noi ricordano il tentativo storico di Giovanni Paolo II, forse il suo grande rammarico che lo accompagnò al termine della sua esistenza terrena, di recarsi a Ur dei Caldei, il luogo di Abramo, il luogo della fondazione delle nostre religioni. Quella delicatezza, quella complessità, quei drammi che si sono succeduti per 2.000 anni purtroppo oggi si stanno trasformando in situazioni molto difficili da governare; tocca però alla politica occuparsene. Se è vero - lo ricordiamo spesso, signora Presidente - che il Corano dice che la parola di Dio è pace e il saluto di un musulmano è *salam aleikum*, la pace sia con voi, se un ebreo si saluta con un suo correligionario con la parola *shalom*, se noi cristiani abbiamo la meravigliosa espressione «*Gloria in excelsis deo et in terra pax

garantire che questo avvenga. È la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che all'articolo 18 recita: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, in pubblico e in privato, la propria religione o il proprio credo, nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti». Queste dichiarazioni esigono reciprocità, esigono il diritto di aprire luoghi di culto, anche luoghi di culto cristiani, in quelle aree dove vige la *Sharia*: vi è il diritto-dovere degli Stati di garantire questi diritti, e della comunità internazionale di pretenderlo dagli Stati che non lo assicurassero. Signora Presidente, quando un cristiano prega non si riferisce a luoghi dell'Occidente, tanto è vero che in fondo anche Roma è una città la cui universalità è difficilmente collocabile storicamente come fatto dell'Occidente. È una città universale per la sua vocazione storica e per la sua bimillenaria natura Ma i cristiani pregano pensando a Nazareth, a Betlemme, a Gerusalemme, non pensano ai luoghi dell'Occidente. Quelli sono luoghi universali, luoghi in cui l'incarnazione di Gesù è stata la concreta testimonianza della vicenda

dalle comunità musulmane in Occidente parole più ferme rispetto a queste situazioni. Ci aspettiamo, se posso usare tale espressione, più coraggio,

civili italiane che partecipavano all'inaugurazione diritto di reciprocità nei Paesi che avevano finanziato la costruzione di quella moschea, per assicurare anche ai cristiani di poter pregare, riunirsi e pacificamente esercitare la propria fede, così come gli ebrei e i credenti di altre religioni. Ecco perché il dibattito di oggi non è solo per

del nostro Parlamento su questi valori, ma è l'occasione per affermare dei principi su cui organizzare e motivare risposte istituzionali e politiche che spettano al nostro Governo, all'Unione europea

quella reticenza di cui parlavo all'inizio e quelle paure che spesso si accompagnano alla denuncia delle persecuzioni nei confronti dei cristiani in troppe parti del mondo diventino azione politica, azione istituzionale, azione di libertà a viso aperto, a partire dalla nostra Repubblica democratica. *(Applausi Presidente, colleghi,

l'impegno che il mio movimento suggerisce, ma che siamo pronti poi a sottoscrivere in modo unitario: un progetto politico che non può essere né di destra né di sinistra né di centro, ma deve essere un progetto di civiltà che il Cristianesimo rappresenta per il nostro mondo.

costituiscono una minoranza, e a valutare l'opportunità di subordinare ogni ulteriore rapporto di carattere politico o economico con tali Paesi all'effettiva tutela, da parte loro, delle parte loro, delle minoranze cristiane presenti sul loro territorio; ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un osservatorio sulla condizione dei cristiani nel mondo, che abbia, tra le altre, funzioni di consulenza al Governo, come quella di valutare il prosieguo delle relazioni diplomatiche, in particolare quelle relative alla cooperazione allo sviluppo che implicano l'erogazione di fondi da parte del bilancio statale, con i Paesi che non garantiscono il rispetto dei diritti delle minoranze cristiane e/o non hanno sottoscritto la Convenzione dei diritti dell'uomo. Avrò poi modo nella dichiarazione di voto di approfondire il mio pensiero personale e quello del mio movimento.

E dice tutto! Effettivamente Maometto è arrivato dopo quasi 650 anni, ed è da lì che è nata tutta la civiltà. La storia è curiosa. Ci propone dei crocevia affascinanti e terribili. Alessandria è il luogo esatto della traduzione del Libro, della cultura ellenistica diventata romana e quindi poi occidentale. Quindi noi stiamo parlando di qualcosa che va difeso. La libertà religiosa, colleghi, è una delle quattro storiche libertà. Abbiamo avuto il coraggio di aggiungerne perché vi sono i nuovi diritti. Ma le storiche libertà sono la libertà d'opinione, religiosa, dal bisogno e dalla paura. C'è tutto qua dentro, perché la libertà religiosa è essenziale, coessenziale alla vita dell'uomo. Si può incatenare un uomo ma non si può incatenare un'idea. Ogni volta che si è voluto distruggere la dignità della persona dalle fondamenta si è cercato di agire sulla sua mente per obnubilarla e per abolirla: basti citare «Se questo è un uomo». Ma poi basti citare cos'è stata l'Armenia e vorrei citare anche i 300.000 sciiti.

discute, come stiamo facendo noi oggi adesso, per far seguire alle parole i fatti, perché la libertà religiosa è la libertà più alta. Chi ha fede ha un Dio con cui parlare, pregare. Chi ha fede deduce che gli altri uomini sono come lui perché figli dello stesso Dio. Che paura si può avere di chi ha nel messaggio del proprio Dio il principio di amare perfino i nemici? È il fondamento della democrazia, perché si dialoga e si fa politica invece di fare la guerra. Quindi, che paura avere anche per coloro che vogliono essere inutilmente laicisti o atei a parole, e che paura invece fanno gli integralisti che piegano invece Dio ai bisogni politici? Di questo si tratta, signora Presidente, colleghi. È il Nord Africa; è proprio da parte di quel mondo da cui viene il Cristianesimo i copti sono la comunità più antica dei cristiani nel Medio Oriente - che ci arrivano messaggi importanti. Lì i cristiani, come per i fedeli di altre religioni in altre parti dell'Oriente, sono utilizzati per rendere esplicito un conflitto politico.

le armi con le quali combattere non sono quelle che impediscono la sopravvivenza del genere umano, ma quelle del diritto internazionale, degli accordi pattizi. A un Governo possiamo chiedere di rispettare i patti.

con un lunghissimo e faticoso processo ai principi condivisi. Da qualche anno, insieme alla Croce rossa ed alla Mezzaluna rossa, c'è anche il *Magen David Adom,* ossia la stella rossa di Davide: siamo arrivati fin lì perché abbiamo cercato di condividere princìpi comuni. Credo che questo Parlamento oggi

i patti che valorizzano i diritti umani più di quelli che valorizzano le transazioni economiche. So che questi ultimi

Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, l'argomento al nostro esame ha certamente una sua attualità, ed alla strage di Alessandria d'Egitto fanno riferimento un po' tutte le mozioni. Ma al di là dell'attualità, le mozioni in discussione cercano di avere una loro profondità e di guardare anche più indietro.

come combustibile con il quale alimentare il cosiddetto scontro di civiltà, ed ha aggiunto due condizioni: la prima è di non partecipare ad accreditare come vero Islam quello aggressivo e fondamentalista; la seconda è non considerare la presenza dei cristiani in Medio Oriente come mero avamposto dell'Occidente. Le due considerazioni del collega Tonini valgono certamente, ma contengono entrambe una loro fortissima carica di ambiguità, e per la stima che ho nei confronti del collega Tonini vorrei contribuire a diradare tale ambiguità. tale ambiguità. Stiamo attenti, collega Tonini. Ricordo un precedente alla mia memoria ben fermo. Eravamo nel 2006, al principio dell'anno, in una sede non sospetta di antioccidentalismo, all'Assemblea di Vienna dell'OSCE. Quel giorno, all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, i Paesi occidentali, gli europei, e anche gli americani, fecero a gara in una competizione in ordine alla quale vorrei parlare di pavidità, ma, siccome ero presente da cronista, dovrei dire di viltà! Consentimmo che un Paese civilissimo come la Danimarca fosse accusato di ogni nefandezza: si parlò di una regina danese che beveva sangue musulmano la mattina al *breakfast*,

è vero che probabilmente i vignettisti danesi erano stati sguaiati e di cattivo gusto, ma quella difesa intransigente della libertà religiosa il collega, e, se mi posso permettere, amico Tonini, ci ha invitato a fare non implica l'abdicazione a considerare la libertà religiosa una fondamentale libertà d'Occidente, quindi una libertà individuale, una libertà con garanzie di reciprocità e quindi non barattabile - è il caso della Danimarca - con la libertà di stampa, con il veto della censura, con la mano legata dietro la schiena nel cosiddetto conflitto di civiltà. Il secondo precedente storico, lo ha ricordato illustrando la mozione del proprio Gruppo il collega Quagliariello, è quello Ma vi siete dimenticati di quell'assassinio di rappresaglia? Perché di rappresaglia? Per la citazione del discorso di Ratisbona di Benedetto XVI. Suor Leonella fu uccisa, barbaramente ammazzata, e ci furono penne occidentali attribuirono le ragioni di quel barbaro assassinio all'imprudenza filologica del Papa, per quella inopportuna citazione di Manuele II Palelologo. mi auguro, come auspicava il senatore Rutelli, che si possa approdare perlomeno a un dispositivo di convergenza, collega Tonini non sono interpretate alla luce delle considerazioni storiche che mi sono permesso di sottoporgli, penso che avremo fatto poca strada nel diradare le ambiguità degli ultimi anni.

si viene uccisi nelle cattedrali, si muore sulla soglia delle chiese, nel mondo di oggi come nei secoli antichi, per il fatto di essere cristiani: l'uomo crocifisso di nuovo ad opera dell'uomo. Ciò che sta accadendo in Egitto, e prima ancora in Iraq, nel Medio Oriente, in Nigeria, in Pakistan e nel Sud Est asiatico, è un tragico segno del tempo che stiamo vivendo, il tempo della paura, della chiusura, del nemico identificato nel diverso, della religione come strumento di scontro, dell'uso politico di Dio. un campo sconfinato, necessario e urgente davanti a noi, quello del dialogo interreligioso, del pluralismo, dell'iniziativa politica per spegnere le tensioni religiose, per prevenirle, per fermare le violenze e il terrorismo. In questo nostro tempo in cui acuto si fa il confronto tra Occidente e Islam, confronto di cui anche la Chiesa cattolica universale è parte, abbiamo non soltanto la responsabilità di denunciare, di comprendere la portata storica del processo in atto e di agire. Democrazia, religioni, pace sono realtà interconnesse e strategiche del nuovo secolo; questa è la sfida, insieme con l'economia globale, per aprire la strada ad una convivenza umana matura, per non ripetere gli orrori del Novecento e dei secoli precedenti e per raccoglierne invece l'eredità evolutiva. Le Carte costituzionali, a partire dalla nostra che all'articolo 19 riconosce a tutti il diritto a professare liberamente la propria fede religiosa, e la Dichiarazione universale dei diritti umani, che all'articolo 18 riconosce sotto tutti i cieli la libertà religiosa come costitutiva della libertà della persona, sono il fondamento per l'uguaglianza di tutti i cittadini all'interno delle nazioni, senza alcuna discriminazione. È questa la base per la stessa legittimazione degli Stati nel contesto internazionale, la cui autorità è messa a rischio dai movimenti di intolleranza e di violenza. L'Italia, allora, si muova in questo solco all'interno dell'Unione europea, nell'ONU e nei rapporti con i Paesi oggi coinvolti in questi avvenimenti e con le aree strategiche teatro delle persecuzioni e delle stragi. Come non vedere che la pace è l'esito, ma anche la condizione per la convivenza tra religioni diverse, come dimostra il Medio Oriente, terra da secoli abitata da cristiani, ebrei e musulmani. La fine della cristianità in Medio Oriente, ha detto il vescovo Audo di Aleppo, sarà una sconfitta anche per i musulmani, perché questo vuol dire la fine dell'antica tradizione di convivenza. La guerra in Iraq a cui noi siamo stati contrari ha rotto quell'equilibrio delicato. Benedetto XVI ha annunciato per quest'anno l'invito, 25 anni dopo l'incontro di Assisi, di capi delle religioni. Vorremmo che fosse il punto di arrivo di un grande cammino condiviso da tutte le comunità del pianeta. La politica ha un compito irrinunciabile con una visione di lungo respiro che noi evochiamo in quest'Aula: intervenire prontamente per costruire la pace con gli strumenti della democrazia, del diritto internazionale e della diplomazia, della cultura

condividono oggi lo sgomento, il dolore per ciò che accade e l'obiettivo di un futuro storico condiviso tra le religioni e le culture diverse. Una convivenza che diventa storia, cultura, comune umanità, pace.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, era il 30 ottobre 2008 quando quest'Aula fu chiamata a votare la mozione sulla persecuzione dei cristiani in India. Oggi, a distanza di due anni, ci riuniamo per fare nuovamente sentire la nostra voce contro la strage avvenuta nella notte di san Silvestro in Egitto. Con tristezza siamo costretti a prendere atto che è cambiato lo scenario geografico, gli autori delle violenze: ieri i fondamentalisti indù, oggi quelli islamici, ma per il resto è tutto uguale. Uguali sono le ragioni di questa cristianofobia divampante, uguale è la mappa luttuosa dei Paesi in cui le minoranze religiose sono offese, umiliate, uccise, costrette all'esodo. Noi tutti, onorevoli senatori, vogliamo sentirci testimoni del valore inalienabile della libertà di religione, ovunque essa avvenga e per qualunque espressione di fede. Ma è dei cristiani perseguitati che oggi dobbiamo parlare, perché sono questi le principali vittime della violenza interreligiosa (ancora una volta di professione cristiana erano le 13 persone rimaste uccise nell'attentato di ieri in Nigeria). Ma è pur giusto che analizziamo quanto accade in un contesto più ampio. Forse questa cristianofobia non si nutre anche del processo di indebolimento identitario e culturale in atto in Europa? In nome di un'Europa pluralista e del relativismo culturale, la civiltà occidentale si è negli ultimi anni mostrata sì comprensiva, accogliente e rispettosa dell'altro, ma purtroppo fino al punto di rinnegare addirittura le proprie radici cristiane, che non hanno potuto trovare neanche diritto di cittadinanza nella Costituzione europea. Ma la difesa della reciprocità, della tolleranza e della convivenza con gli altri popoli non può portaci fino all'abiura della nostra identità, fino ad arrivare a rinnegare le radici della nostra fede. In nome di un laicismo fondamentalista, nel vecchio continente si vogliono eliminare i crocifissi dagli edifici pubblici, mentre in Egitto le donne cristiane sono costrette a portare il velo islamico; in alcuni Paesi europei l'obiezione di coscienza in materia di aborto è sempre più limitata, mentre cresce inesorabilmente la diffidenza verso la religione. di tifoseria per la mia parrocchia, preferisco citare uno stralcio dell'elzeviro scritto ieri dal laicissimo napoletano Raffaele La Capria sul «Corriere della Sera» a proposito della debolezza dell'Occidente: «Noi non ci amiamo più, non consideriamo più con la dovuta sacralità i principi che regolano le nostre società, un senso di colpa e di frustrazione ci accompagna, c'è un sentimento di decadenza inarrestabile che ci colpisce nonostante i traguardi raggiunti dalla scienza, anzi forse proprio a causa di questi è nata un'insoddisfazione che rende le nostre vite prive di quella spiritualità necessaria a sostenerle. Insomma non abbiamo più fiducia in noi stessi, mentre ne occorrerebbe molta per salvaguardare la nostra civiltà che è quella irrinunciabile dei diritti umani» Non possiamo allora che ripartire dalla riscoperta della nostra identità, della nostra eredità culturale greco-romana e giudaico-cristiana che ci ha consegnato una piattaforma comune di diritti e di doveri a partire dalla quale persone di diverse appartenenze, tradizioni, religioni e convinzioni possono lavorare insieme in pace ed uguaglianza. E in fondo mi chiedo che Europa è questo moderno continente che ha promosso e reso possibile la Dichiarazione dei diritti dell'uomo se non è capace di difendere la sacrosanta libertà religiosa. Signora Presidente, onorevoli senatori, sulle festività appena trascorse si è addensata la funerea nube della strage compiuta ad Alessandria d'Egitto. E, sovrapponendosi alle notizie dell'immane carneficina, quanto ci è apparsa stridente l'atmosfera lieta e ovattata del Natale e del Capodanno nelle nostre città! Altrove, infatti, una comunità lontana sulle carte geografiche, ma così prossima per cultura e tradizione religiosa, piange 21 morti e 80 feriti. Il bilancio dell'orrendo attentato avvenuto la notte del 31 dicembre, ordito ed eseguito da menti e mani scellerate, parla di famiglie distrutte e persone uccise La colpa di questi martiri, straziati davanti alla loro chiesa, era quella di professare la religione cattolica, cioè la fede dei loro padri e della propria terra. Lo ribadisco, colleghi senatori, la religione della loro terra. E ricordo una bella espressione di Benedetto XVI in proposito (oggi abbiamo ricordato giustamente in tanti Papa Benedetto XVI). In Medio Oriente, sottolineò il Papa, «i cristiani sono cittadini originari e autentici». Dunque, aggiungo, tali vanno considerati, a dispetto del luogo comune che li vorrebbe quasi dei corpi estranei, delle minoranze occidentalizzate, magari dei residuati del colonialismo. In realtà i Paesi extraeuropei che, dall'altra sponda del mare, si affacciano sul Mediterraneo furono la culla del Cristianesimo (lo ha ricordato bene il senatore Rutelli), Egitto compreso. Qui trovò terreno fertile la prima evangelizzazione che fruttificò lungo i secoli, sino all'invasione maomettana. Risale, infatti, al I secolo la fondazione della Chiesa copta, originata dalla predicazione di san Marco, dove brillò per zelo e dottrina il patriarca san Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa. Nell'arco di due millenni, sotto il duro tallone del conquistatore musulmano, i cristiani d'Egitto hanno strenuamente custodito la propria identità, subendo sistematiche spoliazioni dei beni, rapimenti di fanciulle, uccisioni d'innocenti, inique condanne, angherie innumerevoli e tanto penose da indurre molti alla sofferta scelta dell'emigrazione. Tuttavia i copti rimasti nel loro Paese costituiscono ancora il 10 per cento della popolazione egiziana: una presenza scandalosa agli occhi del fanatismo islamico. scorso, in occasione del tradizionale incontro con i rappresentanti dei Paesi e delle organizzazioni internazionali che intrattengono rapporti diplomatici con la Santa Sede, Benedetto XVI, riferendosi alle stragi di cristiani in Iraq ed Egitto, si è soffermato su quella che ha definito come «urgente necessità per i Governi della regione di adottare, malgrado le difficoltà e le minacce, misure efficaci per la protezione delle minoranze religiose». Ebbene, noi crediamo che della difesa dei cristiani possano e debbano rendersi partecipi gli Stati che, come il nostro, hanno contratto un inestinguibile debito di civiltà nei confronti del cristianesimo. dovere morale ma anche reale, di coscienza e di sostanza, assodata l'esistenza di una lista di circa 200 esponenti della comunità copta che l'estremismo maomettano vuole uccidere, come rivela l'agenzia missionaria AsiaNews; la metà di questi bersagli umani vive - appunto - nei Paesi europei. D'altro canto abbiamo constatato, in occasione del *sit in* dei copti davanti davanti al consolato egiziano di Milano, quanto odio certi islamici nutrano nei confronti dei cristiani egiziani: solo un intervento muscoloso delle forze dell'ordine, a suon di manganellate, ha impedito che chi manifestava solidarietà alle vittime della strage di Alessandria d'Egitto venisse aggredito da gruppi di facinorosi di fede musulmana (sottolineo

parecchie decine di omosessuali ottengono lo *status* di rifugiato o un permesso umanitario per il fatto di non poter manifestare liberamente nei Paesi d'origine certe tendenze sessuali. A questa stregua, quanta considerazione dovremmo mostrare nei confronti di tutti i cristiani copti che quotidianamente rischiano la vita per la fede? Specularmente, quale trattamento riservare ad altri immigrati che abbracciano le credenze degli oppressori? È ammissibile che chi approda nel nostro Paese per sfuggire alla persecuzione religiosa qui incontri i propri aguzzini? Potremmo facilmente dare risposta a tali questioni se certe imposizioni antidiscriminatorie non ci allontanassero spesso dal campo del buonsenso e dell'equità. Si tratta di quel buon senso, come dicevo, che ho sentito echeggiare nelle parole di un amato pastore della Chiesa cattolica, il cardinale Giacomo Biffi,

non è una landa deserta o semidisabitata, senza storia, senza tradizioni vive e vitali, senza una inconfondibile fisionomia culturale e spirituale, da popolare indiscriminatamente, come se non ci fosse un patrimonio tipico di umanesimo e di civiltà che non deve andare perduto. (...) In una prospettiva realistica, andrebbero preferite le popolazioni cattoliche o almeno cristiane». Il cardinale

Ora, il massacro di Alessandria d'Egitto, seguito alle stragi di cristiani in Iraq e alle persecuzioni nel mondo islamico (e penso alla condanna a morte per «blasfemia» per «blasfemia» di Asia Bibi in Pakistan) devono, appunto, indurci a porre con forza il principio della reciprocità all'ordine del giorno dell'azione politica e diplomatica. Concludendo, se si ritiene che, in virtù di regole antidiscriminatorie acriticamente applicate, non sia possibile opporre il rifiuto alle crescenti pretese degli islamici, almeno ci si premuri di esigere che i Paesi d'origine di tali immigrati attuino la parità del trattamento nei confronti delle comunità di cristiani che vivono sul loro suolo. A questo scopo appare auspicabile la costituzione di un organismo intergovernativo a livello europeo, in grado di monitorare costantemente le condizioni di vita delle comunità cristiane nel mondo. E occorre, in modo ancor più necessario, la determinazione dell'Unione europea e dei Governi nazionali a condizionare ogni rapporto di carattere politico ed economico con tali Paesi all'effettiva tutela delle minoranze cristiane presenti sul loro territorio. Crediamo che passi decisi, mossi in questa direzione, raccolgano in maniera concreta l'esortazione del Papa, affinché nella difesa della vita e della libertà dei cristiani seguano finalmente alle parole i fatti.

appartenente all'ultima minoranza cristiana perseguitata sul territorio che oggi costituisce la Repubblica italiana. Per poter sviluppare il mio ragionamento con sufficiente ampiezza, chiedo però di allegare ai Resoconti della seduta

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'analisi dei fatti in politica deve portare a pensare e promuovere possibili soluzioni, se l'analisi è sbagliata il rischio di produrre, nella migliore delle ipotesi, delle terapie inadeguate e, nella più concreta, delle soluzioni sbagliate - quindi anche dannose - è elevato. Se l'analisi dei fatti che ci hanno portato a questo dibattito, a partire dalla morte dei cristiani copti ad Alessandria d'Egitto, è che essi sono il frutto e l'esito di uno «scontro di civiltà», «attacchi e persecuzioni dei cristiani da parte dei musulmani», di «epurazioni», di «pulizia etnica» dei cristiani dal Medio Oriente, di veri e propri nuovi *pogrom* nei confronti delle comunità cristiane, allora parlare - come ha fatto poco fa il senatore Quagliariello - di «cristianofobia» può avere un senso e quindi può sembrare adeguata anche la soluzione, individuata ad esempio dal ministro Frattini, di stipulare accordi in cambio dei diritti dei cristiani nel mondo arabo e musulmano. Ma siamo sicuri che l'analisi sia giusta? Emma Bonino nei giorni scorsi ha tentato di proporne un'altra, diversa, recuperando tra l'altro quella di molti intellettuali arabi, oltre che di donne e di uomini impegnati in associazioni e movimenti della società civile, che ben conoscono quelle realtà. Guardando ad esempio all'Egitto o all'Iraq, per non parlare dei talebani in Afghanistan, l'obiettivo che l'Islam combattente intende perseguire con l'arma del terrore è un altro: liquidare l'Islam dialogante, quello più ragionevole. Allora, più che davanti ad uno scontro di civiltà o a una guerra di religione, ci troveremmo davanti ad uno scontro interno tra l'Islam combattente e quello più «ragionevole», quello più secolarizzato, quello più dialogante con l'Occidente. Che una delle conseguenze di questo scontro in atto, all'interno però dell'Islam, sia una situazione di grande instabilità, di paura, che può produrre anche degli esodi di quanti si sentano minacciati, è un fatto grave e incontestabile. Ma non è questa la ragione, la motivazione degli attacchi: il discorso vale per l'Egitto, ma a ben vedere, anche per l'Iraq. Gli islamisti combattenti fanno anche dei calcoli politici; il loro scopo non è il terrore per il terrore. Costoro colpiscono nelle zone «fragili» - è il caso dell'Iraq - o in zone consolidate che stanno però attraversando una fase di transizione complessa: questo è il caso dell'Egitto. Allora ecco perché in Egitto, per esempio, l'obiettivo vero e strategico dei terroristi e dei loro mandanti non sono tanto i copti, i cristiani, ma è la classe dirigente araba, a cominciare da Hosni Mubarak, considerato un «fantoccio nelle un «fantoccio nelle mani dell'Occidente». Insomma, più che uno scontro di civiltà tra Occidente e Oriente, si tratta di una duplice resa dei conti all'interno delle all'interno delle varie anime politiche ed identitarie dell'Islam. Restando in Egitto, la prima sfida è quindi quella tra gli islamisti islamisti militanti, i jihadisti, e la *leadership* araba di Mubarak, più secolarizzata e dialogante con l'Occidente. C'è poi un'altra sfida, non meno significativa, che riguarda l'egemonia del variegato arcipelago fondamentalista.

soluzioni aderenti alle realtà in questione, i vecchi *cliché* della contrapposizione tra la civiltà islamica e quella cristiana, rischiando di fare così proprio il gioco di chi sta minando la classe dirigente araba moderata per sostituirla con una ben più integralista.

come a dire a tutti gli abitanti della Terra, eccetto quelli dei Paesi democratici. Quando si tentò di inserire un riconoscimento nel Trattato per la Costituzione europea delle comuni radici giudaico-cristiane, alcuni Paesi posero Paesi hanno preso posizione per la tutela dei cristiani perseguitati. La ragione è piuttosto evidente, dal momento che su quelle radici si innesta un diritto fondamentale dell'uomo, quello che esprime il suo bisogno di spiritualità e che oggi, più che mai, è essenziale per la pace. È chiaro che qualsiasi scelta di coscienza, da quella religiosa a quella di pensiero o politica, deve essere rispettata e tutelata, ma non possiamo agire da soli, dobbiamo lavorare tutti insieme. L'Unione europea deve sentirsi coinvolta per difendere le sue radici, non solo con manifestazioni di sdegno per gli eventi di questi giorni, ma anche con un impegno comune per reclamare il rispetto della libertà religiosa di tutti, quale diritto inalienabile di ogni uomo, un diritto proprio delle persone, non concesso dagli Stati, ma patrimonio dell'individuo. È indispensabile che i Paesi esigano a livello internazionale il rispetto della libertà di culto e la pretendano in termini di reciprocità. motivo occorre perseguire, in sede ONU, la piena applicazione dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata nel 1948, sulla libertà di religione. Quanto ha fatto l'Italia in occasione della 65a Assemblea generale dell'ONU, sul tema della tolleranza e della libertà religiosa, rappresenta già un passo in avanti importante, ma non basta. Bisogna abbandonare in sede internazionale un altro concetto terribile, che è quello della diffamazione religiosa, che serve solo da pretesto, specie agli Stati islamici, per perseguitare le minoranze cristiane, poiché i diritti dell'uomo debbono proteggere gli individui e non alcune fedi religiose. La battaglia istituzionale quale la diplomazia italiana si era impegnata a nome delle minoranze religiose non è finita e richiede di essere ripresa con determinazione.

Bisogna tutelare la possibilità di esprimere la propria fede non solo nel privato, ma anche nel pubblico. Affermare la libertà religiosa non vuol dire far diventare lo Stato confessionale: vuol dire riconoscere agli individui il diritto di poter professare liberamente il proprio credo. Se crediamo davvero che la libertà religiosa non possa dirsi patrimonio esclusivo dei credenti ma dell'intera condizione umana, in quanto sintesi di tutte le libertà fondamentali da cui uno Stato di diritto non può prescindere, allora dobbiamo trovare anche in quest'Aula quella unità di intenti che la gravità del problema che stiamo trattando richiede. *(Applausi

di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto(...)». Credo siano queste parole eloquenti che è importante ricordare per fa riemergere nelle nostre memorie il principio che ha ispirato detto assioma. Libertà religiosa, democrazia e pace rappresentano un trittico, tre grandi valori inscindibili, nel quale nessun elemento può esistere senza l'altro.

Peccato che ciò che per noi è considerato scontato per altri Paesi non lo sia affatto e peccato che, solo a seguito dei numerosi episodi di violenza perpetrati in Medio Oriente, oggi, finalmente, le nostre coscienze siano riuscite a risvegliarsi, a dire no con coraggio a chi viola un sacrosanto diritto di libertà: professare la propria fede. Non ci saremmo mai immaginati di assistere ad una così tale ferocia contro chi, condannato perché crede, è stato colpito, messo a tacere, considerato alla stregua di un nemico di Stato. Stato. Sono parole e concetti inauditi. Non mi sarei mai immaginata di dover vivere e discutere di questo all'interno del nostro Parlamento. Negando la libertà religiosa, che è elemento essenziale della democrazia, neghiamo i principi stessi della democrazia. Si tratta di una contraddizione che ci impone una riflessione attenta. In fondo, perché noi sosteniamo che la libertà religiosa è la premessa fondamentale per la democrazia e per la pace? Perché

È qualcosa di fondante dell'essere umano, e questo vale per i credenti, ma anche per i non credenti, vale per tutti gli uomini, per tutte le persone umane. Con amarezza oggi ci rendiamo conto che ciò che abbiamo dato per scontato non lo è. E forse ci siamo spesi troppo ad elaborare i fondamenti filosofici del concetto di libertà religiosa,

dobbiamo assumerci - come hanno detto molti colleghi - degli impegni nell'agenda della politica estera e far sì che il tema della libertà religiosa - abbasso il tono di voce diventi prioritario nelle relazioni internazionali all'interno degli organismi internazionali. Concludo ricordando la regola d'oro, che primeggia nelle relazioni umane,

Cristianamente è la regola dell'amore, laicamente questa è la regola della fraternità universale. È la regola del rispetto, la regola che ci fa dire la libertà religiosa è un principio irrinunciabile e imprescindibile di tutte le relazioni internazionali, oggi più di ieri; è un dovere del Parlamento, e io mi auguro che approveremo tutti lo stesso dispositivo per trasmettere un segnale positivo

Noi però dobbiamo contribuire, grazie a questa unità di fondo, a rafforzare una linea che potremmo riassumere in queste fondamentali e semplici affermazioni: più diplomazia, più politica, più cultura. Dopo la Guerra fredda, chiuso quel lungo periodo di tensioni abbiamo avuto anche in Occidente l'illusione che l'approccio ai grandi problemi del mondo fosse reso più semplice proprio dal fatto che la divisione intervenuta dopo la Seconda guerra mondiale non c'era più. Invece, sono sorti altri problemi, e dobbiamo avere la capacità di recuperare questo senso profondo della diplomazia, della politica e della cultura. È stato già detto nell'intervento svolto in precedenza dal senatore, amico e collega Tonini, che i copti non sono cristiani che appartengono ad una Nazione per caso: sono degli egiziani. Ma io vorrei aggiungere, se mi è consentito, una semplice sottolineatura. Si tratta di una confessione

rivendica una diversa dottrina: sostanzialmente, questa dottrina contestava il Credo che poi è stato assunto dalla Chiesa romana. Con ciò intendo dire che si tratta di cristiani

del Cristianesimo occidentale nel Medio Oriente, in questo caso in Egitto. Sono una comunità autonoma che, nella lontana storia, ha preso le distanze e si è contrapposta a Roma. Ciò significa che, comprendendo la complessità di questi problemi,

di una Nazione, di uno Stato che conosce i problemi interni esistenti tra la comunità musulmana, prevalente, e la comunità cristiana, minoritaria.

produce l'affievolimento di quel concetto, di quella concezione e ne chiede un'innovazione ed una rivisitazione. Facciamolo, dando una spinta unitaria come Parlamento italiano.

che è stata protagonista della nostra storia occidentale, ma una più ampia e importante libertà: la libertà di credere, di vivere ed esprimersi in un mondo in cui pace e tolleranza sono valori indiscussi. È di ieri la notizia di un cristiano ucciso e di altri quattro feriti in un attentato su un treno, nel Sud dell'Egitto. dell'ennesimo attentato, dopo le vere e proprie carneficine che nella notte di Natale hanno visto la morte di almeno 80 persone negli attentati e negli scontri tra cristiani e musulmani nella Nigeria centrale. Ma non è solo in Africa che i cristiani sembrano soffocati da episodi di violenza legati ad estremismi più o meno diffusi. Il rapporto sulla libertà religiosa nel mondo 2010, presentato ogni due anni dall'organizzazione cattolica internazionale Aiuto alla Chiesa che soffre (ACS), rivela che il numero dei cristiani perseguitati nel mondo è di 200 milioni, e quello dei discriminati per la loro religione di 150 milioni. Papa Benedetto XVI, alla vigilia della beatificazione del cardinale John Henry Newman, ha detto: «Nella nostra epoca il prezzo da pagare per la fedeltà al Vangelo non è tanto quello di essere impiccati, affogati e squartati, ma spesso implica l'essere additati come irrilevanti, ridicolizzati o fatti segno di parodia». Il peggioramento della situazione è dovuto soprattutto a una maggiore radicalizzazìone del fondamentalismo islamico, che colpisce non solo i cristiani, ma tutti coloro che non la pensano come i fondamentalisti. Dove non esiste la libertà religiosa non esiste la libertà democratica. Infatti, la libertà di religione non è solo uno dei diritti tra gli altri: è, in è, in un certo senso, la sintesi di tutti i diritti umani. Giovanni Paolo II prima e Benedetto XVI poi hanno affermato ed affermano che la libertà di religione è la base di tutti i diritti, la cartina di tornasole che verifica se davvero in una società vi è libertà. Soffocare la libertà religiosa vuol dire soffocare le libertà civili di un gruppo, che sono la libertà di coscienza, di espressione e di stampa, di associazione. Le limitazioni alla libertà religiosa divengono di fatto limitazioni delle proprie libertà civili di espressione, di stampa, pubblicazione e diffusione; di associazione; di movimento. Si va dal Myanmar, con la sanguinosa repressione dei monaci buddisti, alla Corea del Nord dove è vietato praticare la fede e dove continua a non esserci

Paesi come Cina, Laos, Vietnam, Nord Corea soffrono o addirittura perseguitano la Chiesa cattolica, le Chiese protestanti domestiche, il buddismo, tutte le religioni. La verità è che l'intolleranza religiosa dei nostri tempi è spesso frutto di una netta contrapposizione politica nei confronti del Cristianesimo considerato espressione della cultura occidentale, europea e nord americana. Da parte nostra, da parte cioè dell'Europa, del Nord America e di Israele, è fondamentale la diffusione della tolleranza, del pluralismo tanto politico che religioso. La storia della nostra Europa ha segnato pagine e pagine di conflitti che hanno preceduto la riforma protestante, la nascita del Calvinismo e del Luteranesimo in antitesi al potere dei Papi. Nel Medio Evo, con la lotta per le investiture e gli scontri epocali tra Impero e Papato, si è sviluppata la cultura di convivenza tra religione e autorità politica, in definitiva tra fede e laicato. Le violenze contro la libertà religiosa sono anzitutto attentati contro le persone, ma sono anche attentati contro la società e il progresso civile, sociale ed economico di un Paese. Chi opprime o soffoca la libertà religiosa di fatto sceglie di tenere in condizioni di sottosviluppo il suo popolo. Quello della distruzione delle scuole, per esempio, è un elemento di persecuzione che è ormai quasi un *trend*: in Cina, a Hong Kong, in Indonesia, in Nepal. Non si vuole in questo caso imbavagliare la fede di una comunità: si vuole distruggere la possibile influenza sociale delle religioni, in particolare di quella cristiana. Scuola significa infatti lotta all'analfabetismo, apprendimento di un mestiere, conseguimento di una laurea, educazione, carriera, trasformazione sociale, libertà. Si distrugge quindi non solo per uccidere la fede, ma anche per impoverire, per frustrare il popolo, per avere meno prospettive sociali. In Iraq la persecuzione contro i cristiani va di pari passo con l'eliminazione dell'intellighenzia irachena. La violenza sunnita e sciita sta infatti colpendo anche anche gli intellettuali e i professori universitari: fisici, ingegneri, giornalisti cosiddetti musulmani moderati, che aprendosi al dialogo con altre culture, rischiano di "inquinare" la purità islamica fondamentalista. Da questo punto di vista, l'uccisione, i rapimenti di intellettuali e scienziati in Iraq stanno impoverendo la Nazione e la stanno condannando al sottosviluppo, come e più che la guerra e l'insicurezza. La conclusione è che il potere che soffoca la libertà religiosa pone le basi per la distruzione della società: nei Paesi islamici, perché vi sarà una crescita di fondamentalismo; nei Paesi atei, perché la mancanza di libertà religiosa crea un conflitto sociale sempre più intenso. Senza dignità dell'uomo garantita dalla dimensione religiosa e senza solidarietà sociale, il progresso tecnico tecnico crea ingiustizie, divisioni e conflitti. Si potrebbe obiettare che Cina, India, Maldive, Vietnam, sebbene soffochino la libertà religiosa, sono Paesi ormai ad avanzatissimo sviluppo. In realtà, la violenza sulle religioni è segno di un profondo squilibrio presente nelle loro società, che mette in crisi la qualità umana di tale sviluppo. Analizziamo, ad esempio, il prezzo pagato dalla Cina per lo sviluppo: morti in miniera, disoccupati, pensionati, giovani disperati e suicidi. In Cina, perfino l'alfabetizzazione, l'orgoglio di Mao, è divenuto un bene di lusso: almeno l'80 per cento dei figli dei contadini lascia la scuola dell'obbligo per andare nelle città a lavorare come disperati migranti. Tali squilibri ed ingiustizie nascono dalla mancanza di libertà religiosa, dall'emarginazione della dimensione religiosa nella società. Ricordiamo Benedetto XVI, che nella sua ultima enciclica «*Caritas in veritate*» ha sottolineato che: «Dio è il garante del vero sviluppo dell'uomo», per cui, «la promozione programmata programmata dell'indifferenza religiosa o dell'ateismo pratico da parte di molti Paesi contrasta con le necessità dello sviluppo dei popoli, sottraendo loro risorse spirituali e umane». Senza la libertà religiosa, il super sviluppo di tanti Paesi asiatici, rimane afflitto dal sottosviluppo morale che danneggia lo sviluppo autentico. Nella nostra mozione, la proposta per la convocazione, in sede ONU, di una conferenza internazionale sulla libertà religiosa vuole impegnare i diversi Stati nella prevenzione e nel contrasto del fanatismo e dell'intolleranza religiosa. È estremamente positiva la notizia di oggi che riguarda il superamento del *quorum* del 60 per cento dei voti nel *referendum* per l'indipendenza del Sudan meridionale. Si tratterà di vigilare attentamente per garantire la secessione del Nord islamico e la libertà religiosa di circa quattro milioni di cristiani e animisti. e animisti. Si può affermare che le violazioni alla libertà religiosa avvengono sempre più per motivi di potere e in disprezzo allo sviluppo umano e sociale dell'uomo. In passato, erano molto più frequenti le motivazioni di quel fondamentalismo fanatico che vuole annientare le altre comunità confessionali: il rifiuto di religioni (come il Cristianesimo) legate a un passato coloniale; le motivazioni ideologiche marxiste, che volevano distruggere le religioni considerate come l'oppio dei popoli. Ora invece è chiaro che la lotta contro le religioni è una lotta contro la libertà, per salvare il potere e gli affari delle oligarchie che detengono il potere. Giovanni Paolo II richiamava tutti alla responsabilità di proclamare i valori delle religioni, mai in termini di contrapposizione, ma sempre di dialogo: «Non si uccide in nome di Dio! Chi uccide con atti terroristici coltiva sentimenti di disprezzo verso l'umanità, manifestando disperazione nei confronti della vita e del futuro. Pretendere di imporre ad altri con la violenza quella che si ritiene essere la verità, significa violare la dignità dell'essere umano e, in definitiva, fare oltraggio a Dio, di cui egli è immagine. A ben guardare, il terrorismo strumentalizza non solo l'uomo, ma anche Dio, finendo per farne un idolo di cui si serve per i propri scopi». i propri scopi». In conclusione, dobbiamo tenere ben presente che gli episodi di intolleranza e di chiusura verso la religione cristiana, che avvengono in molte parti del mondo, non devono farci arroccare nella cieca difesa dell'identità, minacciata dalla paura della diversità.

quale riflessione sia possibile fare oltre alle domande che gli atti persecutori e violenti che hanno segnato questi giorni e queste ore pongono al tempo nel senso della storia, allo spazio nel senso dei luoghi, alle moltitudini nel senso dei popoli, e a ciascuno di noi, poiché credo sia indifferente a fatti forse lontani per quanto riguarda gli spazi, ma certamente non lontani per quanto riguarda il sentire. Il cristiano è un uomo imbarazzante, soprattutto quando si riunisce in quelle comunità necessarie per proferire le proprie parole e la propria religione. È un uomo imbarazzante perché è un soldato di una rivoluzione incomprensibile: la conversione quotidiana, che è un'esperienza non privata, un'esperienza intima ma non privata, anzi, più è intima e meno è privata, più è intima e più ha necessità di essere pubblica e diventa cosa politica. Un bellissimo film che in questi giorni forse si può ancora vedere in qualche sala e che si intitola «Uomini di Dio» racconta come in un monastero nelle montagne dell'Algeria, nei primi anni monaci trappisti furono trucidati semplicemente perché erano lì, perché quel monastero rappresentava una realtà politica, proprio in quanto si viveva una dimensione profondamente intima. Il cristiano tenta di essere un uomo libero che grida la libertà per tutti, anche per quelli che professano credi e religioni diverse, ed è per questo che diventa talvolta incomprensibile. È un uomo che ha la convinzione e la certezza che ci sono cose per cui vale la pena spendere la vita o addirittura darla, offrirla fino all'estrema conseguenza, e in alcuni luoghi del mondo andare in Chiesa è un atto di coraggio che mette a repentaglio la propria vita. Così, questo uomo imbarazzante usa uno strumento che direi scandaloso, bizzarro,

sappiamo dovremo concludere con una visione comune, con un voto che sottolinei come anche questo Senato, come la Camera ha fatto oggi, ha su tale materia una posizione unitaria), ma in termini diversi.

Eppure, so che la reciprocità deve essere presente in un'agenda politica adulta, e certamente non mi dissocio da tale necessità. C'è bisogno di Europa, lo dicono tutte le mozioni.

davvero debba ricostituire quel sentimento per cui la conversione quotidiana è stata il fondamento di questa Europa. Penso che occorra evitare che la persecuzione di quei luoghi si traduca in un pregiudizio all'interno della più civilizzata Europa, che vorrebbe confinare a quella dimensione privata, che non è possibile per un cristiano, l'espressione della propria fede. La libertà religiosa è una autentica via verso la pace: lo afferma proprio il Papa, e certamente capiamo che si tratta di un passaggio che non può non interessare ognuno di noi. C'è qualcosa che ciascuno di noi può fare oltre a sostenere, come facciamo in questo momento, momento, una mozione unitaria, un atto che richiami l'Europa e le organizzazioni internazionali. Sì, c'è qualcosa che penso possiamo fare: un'autentica arma della pace, la definisce il Pontefice, con una missione storica e profetica, quella di cambiare e rendere migliore il mondo. Un pezzetto davvero ciascuno di noi lo può fare. Uno studente molto impetuoso e ben animato un giorno entrò nella stanza di San Francesco di Sales e gli chiese: «Padre, che cosa posso fare per la pace nel mondo?».

il senatore Rutelli ha richiamato poc'anzi la Dichiarazione dell'ONU del 1948 che costituisce uno standard vincolante per tutti i Paesi membri dell'ONU, nessuno escluso: una concezione piena della libertà religiosa, non di semplice tolleranza, che prevede anche il punto delicato ma chiave della possibilità per la singola persona di cambiare religione.

che segnò l'inizio della nuova storia di libertà religiosa, e cioè la seduta dell'Assemblea costituente del 25 marzo 1947, i cui atti ho inviato come regalo di Natale per e-*mail* a tutti i colleghi,

De Gasperi afferma tre principi che vorrei ricordare, il primo dei quali è il fondamento stesso della Dichiarazione dell'ONU: lo Stato non può avere il controllo delle coscienze. La libertà di coscienza e religione è un sacrario della senatrice Baio)*. Dice De Gasperi: «Anche coloro che si arrestano sulla soglia dei misteri della fede e si preoccupano sostanzialmente della morale sociale sentono (e qui è una questione di esperienza di tutti gli uomini che sono al Governo) che lo Stato non ha la forza, l'autorità di affermare e dirigere la coscienza della singola persona». Nessuno Stato ha questo diritto. Nessuno Stato può con la coercizione violare la coscienza personale. Il secondo passaggio riguarda il Trattato di pace che richiede all'Italia di impiantare un sistema di libertà di coscienza e religione in precedenza negato. Ciò ci richiama alla tutela universale dei diritti umani, al superamento della sovranità assoluta dello Stato. dello Stato. Infine, De Gasperi conclude con il fondamento storico concreto dell'affermazione di questa libertà: la tragedia comune delle guerre che derivava dalla coercizione sulla coscienza personale e dalla sovranità assoluta degli Stati. Dice De Gasperi: «in certi conventi erano ammassati e nascosti cattolici, protestanti ed ebrei insieme. Si trovavano uniti la sera, nei momenti tragici e nei momenti delle minacce. Questa è la nostra forza: se in Italia creeremo una norma di tolleranza per tutti, ma soprattutto una norma in cui si riconosca questa paternità comune che ci protegge e che protegga soprattutto la Nazione italiana». E allora noi insistiamo perché l'ONU si faccia carico di garantire gli standard che la sua Dichiarazione impone a tutti gli Stati membri. Quanto a noi, dobbiamo insistere per questo, ma per inciso dobbiamo riconoscere che c'è qualche piccolo passo che dobbiamo compiere anche noi. In Commissione affari costituzionali ci sono intese siglate dall'attuale Governo.

La strage dei cristiani in Egitto che ha aperto il 2011 proietta una luce pericolosa su questo nuovo anno mettendo però anche in evidenza la debolezza interiore dell'Europa e dell'Occidente, succubi del relativismo religioso, del laicismo imperante che continua ad aprire, in forma del tutto arbitraria, le porte alle frange più pericolose, arroganti e violente dell'Islam. Ritengo che le istituzioni europee fino ad oggi non abbiano saputo reagire alle numerose offese, ingiurie e spesso oscenità perpetrate contro la religione cristiana, dimostrando così che non abbiamo più la certezza di chi siamo e che preferiamo presentarci dovunque senza radici: nella fede, nei valori e nell'identità. Tale comportamento ci fa percepire, proprio da quelle frange estremiste di una certa parte dell'Islam, come un territorio di conquista. Nella mozione che avevo presentato non molto tempo fa, sottolineavo il fatto che il degrado di tutto l'Occidente, al quale non è assolutamente immune l'Europa, immune l'Europa, sia frutto dell'errata convinzione che l'unico processo per l'integrazione degli immigrati passa attraverso la strada di un multiculturalismo anticristiano; i danni di tale decisione li subiamo ormai quotidianamente. Basti pensare al no all'affissione del crocifisso nei luoghi pubblici, al no al presepe nelle scuole

Il XX secolo ha visto il più grande massacro di cristiani che si sia mai verificato nella storia e, a tutt'oggi, il Cristianesimo è di gran lunga la religione più perseguitata al mondo. L'inasprimento delle persecuzioni contro i cristiani è ormai senza confini: colpisce i Paesi asiatici, africani, sudamericani, ma in modo ancora più violento e subdolo quelli mediorientali ed europei. È ora di dire basta; è ora che anche i nostri politici che si professano «laici cristiani impegnati» lo dimostrino con i fatti; è ora che l'Occidente e l'Europa, in particolare, abbiano il coraggio di reagire e di difendere senza alcuna esitazione le nostre radici cristiane, così come il principio della libertà religiosa, quale diritto unico ed inviolabile per tutti, garantendo ai cristiani di tutto il mondo, anche là dove sono minoranza, di pregare e vivere in piena sicurezza senza subire alcun genere di violenza o sopruso che li costringe, sempre più spesso, ad abbandonare la propria casa ed il proprio Paese. Il Cristianesimo è la religione del dialogo e della tolleranza, ma anche, e soprattutto, del rispetto per la persona e dell'amore per il prossimo; principi, questi, da sempre alla base di tutte le Costituzioni occidentali. penso che anche quest'Aula debba chiedere a gran voce al Governo italiano, ma attraverso un impegno di tutti quanti noi, di continuare a difendere il rispetto delle nostre tradizioni e della nostra religione - come bene ha fatto in questi mesi il ministro Frattini - per garantire alle nuove generazioni la possibilità di vivere in una società democratica, libera, dove si possa professare ogni religione, la propria religione,

a nome del Governo, ringrazio tutte le forze politiche presenti nell'Assemblea del Senato per il confronto estremamente approfondito ed importante che si è svolto in quest'Aula, ma soprattutto per la conclusione a cui si è arrivati, cioè un documento unitario e - cosa ancor più importante, che tengo a ribadire - un documento unitario che risponde, nella sua quasi totalità, totalità, al testo che è stato approvato questa mattina, egualmente in maniera unitaria, alla Camera dei deputati. Credo che questa sia la dimostrazione del valore che il Parlamento italiano e le forze politiche attribuiscono ad un tema così delicato. attacchi di cui sono state oggetto le comunità cristiane nel mondo rappresentano, per noi, un segnale di una preoccupante tendenza che mette in pericolo i principi della libertà di religione e la stessa esistenza di queste comunità religiose. Si tratta di una grave minaccia - come è stato evidenziato più volte - per i principi e le libertà fondamentali che dovrebbero costituire la base della convivenza pacifica e dell'ordine internazionale.

- per quel che ci riguarda - fossero una delle principali azioni politiche dell'Unione europea. Nei giorni scorsi il Governo, attraverso il ministro Frattini, si è fatto promotore, con diversi partner dell'Unione europea, di un'iniziativa per iscrivere l'argomento della libertà religiosa e persecuzione dei cristiani nel mondo a pieno titolo nell'agenda del Consiglio affari esteri dell'Unione europea che si svolgerà il 31 gennaio A questo fine, il 5 gennaio è stata inviata all'alto rappresentante Catherine Ashton una lettera firmata congiuntamente

Ricordo che i Ministri ungherese e polacco hanno firmato rappresentando essi le due Presidenze che si succederanno nel 2011. Riteniamo che questo dossier debba meritare la massima attenzione, sia a livello politico sia da parte delle strutture del Servizio europeo di azione esterna e che esso debba rappresentare una delle grandi priorità dell'agenda comune europea. Se le minoranze cristiane vengono perseguitate nel mondo, l'Europa deve parlare. Tali preoccupazioni erano, peraltro, alla base di diverse iniziative intraprese nel recente passato dall'Italia in sede europea ed internazionale, anche grazie a specifiche sollecitazioni del Parlamento italiano. La difesa della libertà religiosa e di culto e la tutela degli appartenenti a minoranze religiose costituiscono da tempo una delle priorità della politica estera italiana nel campo dei diritti umani. La discriminazione basata sulla religione (che non è limitata ad una specifica confessione né ad una specifica regione del mondo, ma che negli ultimi tempi ha colpito in modo particolarmente efferato le minoranze cristiane) rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani. Già alla fine del 2009, prendendo spunto dai numerosi attacchi avvenuti in diversi Paesi contro le minoranze religiose - in particolare quelle cristiane l'Italia aveva promosso l'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, di Conclusioni *ad hoc* sulla libertà di religione e successivamente, nel giugno 2010, di un Piano d'azione in tal senso. Al Consiglio affari esteri dell'Unione europea del 13 dicembre scorso si è inoltre deciso, a seguito di un'iniziativa presa congiuntamente da Italia e Austria e sostenuta da altri partner, che l'Unione europea elaborerà periodicamente un rapporto sullo stato della libertà religiosa nel mondo. Da ultimo (il 21 dicembre 2010) è stato elaborato dall'Unione europea un documento di lavoro intitolato «Messaggi chiave: linea da assumere su libertà di religione e di credo». Tale documento impegna le delegazioni dell'Unione europea nei Paesi terzi sui punti essenziali che devono caratterizzare la posizione europea in materia di libertà di religione. Non stiamo parlando del punto di arrivo di questo dibattito, ma, vogliamo sottolinearlo, solo di una base di partenza di un processo che dovrà portare l'Unione europea ad un maggiore e più efficace coinvolgimento su questo dossier, sia sul piano bilaterale dei rapporti con i Paesi terzi che nell'ambito dei diversi fori multilaterali competenti (ONU, G8, OSCE e Consiglio d'Europa). Tra le possibili misure da sviluppare, voglio ricordare al Parlamento le seguenti iniziative: inserire in modo sistematico nell'agenda di ogni incontro di dialogo politico dell'Alto Rappresentante dell'Unione europea con i Paesi terzi il tema dei diritti umani e, in particolare, quello della libertà religiosa; sviluppare tra i programmi di cooperazione dell'Unione europea con i Paesi terzi una particolare attenzione a quelli relativi all'educazione, al rispetto dei diritti umani e al dialogo interculturale e interreligioso; promuovere la cooperazione tra Unione europea e Stati della sponda Sud del Mediterraneo in materia di antiterrorismo, con riferimento specifico agli attacchi terroristici contro individui o gruppi di individui inermi, comprese le comunità religiose; e sollecitare i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo ad affrontare gli attuali difficili momenti in maniera coerente e democraticamente accettabile.

«contro il terrorismo e a favore della convivenza civile e religiosa tra i popoli», intendendo che «hanno avuto luogo atti ricorrenti di violenza contro cristiani copti», ma in un quadro - ripeto - di azione governativa che noi riteniamo accettabile. l'Unione europea deve sollecitare congiuntamente i competenti organi dell'ONU, come l'Alto Commissario per i diritti umani e il Relatore speciale per le libertà religiose, affinché rivolgano la loro principale attenzione alla questione della persecuzione delle minoranze cristiane. Per quel che riguarda l'ONU, desidero

Ciò è avvenuto anche grazie all'azione dell'Italia, che ha spinto perché si arrivasse all'approvazione per consenso della risoluzione, richiamando l'aumento degli specifici episodi di violenza contro gli appartenenti a minoranze religiose e il dovere di ogni Stato aderente all'ONU di esercitare la massima vigilanza per prevenirli e punirne i responsabili. Va anche detto, e non va nascosto a questo Parlamento, che nell'ambito delle Nazioni Unite il negoziato su questi argomenti è sempre molto complesso, sia perché diversi Paesi tendono a subordinare il loro consenso all'introduzione di elementi che noi consideriamo restrittivi e contrari ad esempio, l'eliminazione di riferimenti troppo espliciti al diritto di cambiare religione) sia perché questa iniziativa si collega a quella, portata avanti dai Paesi della Conferenza islamica, sulla «diffamazione delle religioni», che presenta invece numerosi aspetti problematici. Sostanzialmente, secondo i Paesi islamici esiste un vuoto normativo da colmare per tutelare i credenti da forme di attacco e di irrisione della religione islamica e della sua simbologia. Abbiamo sempre risposto, contrariamente all'affermazione dei Paesi della Conferenza islamica, che la diffamazione delle religioni non è un concetto riconducibile al sistema di tutela internazionale dei diritti umani, perché essa può essere usata per limitare la libertà di espressione e di religione. Per questo appare preferibile, secondo il Governo italiano, concentrarsi nel dare attuazione ai numerosi strumenti giuridici e politici esistenti in ambito ONU piuttosto che pensare a iniziative completamente nuove. proposito la Dichiarazione ONU sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione o sul credo, documento fondamentale per la tutela della libertà religiosa, di cui alla fine del 2011 ricorrerà il trentennale. L'Italia sostiene inoltre iniziative di dialogo nell'ambito dell'Alleanza delle Civiltà: rimaniamo convinti che, nell'era della globalizzazione, la promozione della conoscenza e del rispetto reciproco tra i popoli di culture diverse sia uno degli strumenti essenziali dell'azione politica che deve essere svolta da parte del Governo italiano. Sempre sul versante degli strumenti multilaterali, va tutelata la figura e l'indipendenza del Relatore speciale per le libertà religiose, il cui compito consiste nel compiere visite nei vari Paesi, redigere rapporti contenenti raccomandazioni agli Stati per migliorare la tutela della libertà, ed esprimersi attraverso dichiarazioni pubbliche in caso di eventi o situazioni preoccupanti. di un'azione di monitoraggio che, a giudizio del Governo italiano, va rafforzata, resa efficace, ma soprattutto visibile, anche attraverso un più attivo sostegno alla sua attività da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

dichiarazione - a monitorare gli esiti del *referendum* in corso nel Sud del Sudan, veniamo sollecitati a svolgere il nostro doveroso ruolo. Per essere ancora più concreto - e mi rivolgo soprattutto al senatore Rutelli -credo che noi abbiamo di fronte una una necessità che si collega perfettamente alla richiesta che qui viene formulata. Come voi sapete, il *referendum* sarà valido se ci sarà un 60 per cento di partecipanti al voto. Il *referendum* sta andando molto bene, ma siamo ancora al 25 per cento, anche se ci

di Abyei. Se il senatore Rutelli è d'accordo, credo che l'interpretazione pragmatica e concreta della sua proposta impegni il Governo italiano ad essere molto vivo e vigile in questi sei mesi,

noi di Futuro e Libertà riteniamo molto importante quest'ordine del giorno, innanzitutto perché recupera su un tema così delicato e strategico l'unitarietà del Parlamento e poi perché chiama in causa direttamente l'Europa. La libertà religiosa è all'origine dell'Europa, all'origine dell'identità europea, e il Cristianesimo ha dato un contenuto decisivo alla costruzione di questa libertà religiosa. È proprio con la testimonianza ancora una volta di martiri, sempre cristiani, dei martiri delle persecuzioni dell'Impero romano, che si afferma per la prima volta nella storia il diritto di esercitare il culto che si desidera. Tertulliano definisce di libertà naturale per ciascuno praticare il culto secondo quanto egli crede né - dice sempre Tertulliano - compete alla religione costringere alla religione. L'Editto di Costantino del 313 dopo Cristo è la prima Carta costituzionale ‑ passatemi questo termine - nella quale si afferma la libertà per ciascuno, per ogni uomo, di praticare il proprio culto, fosse esso

Occidente - c'è la testimonianza dei padri pellegrini che cercavano una nuova patria dove poter professare liberamente la propria fede. La laicità dello Stato, d'altro canto, si accompagna alla libertà religiosa e ancora una volta chiama in causa direttamente il Cristianesimo: «Date a Cesare ciò che è di Cesare. Date a Dio ciò che è di Dio». lo Stato laico essere cristiani, ebrei e musulmani è del tutto indifferente perché ogni persona ha eguali diritti e le istituzioni non possono imporre a nessuno un credo. Ognuno sceglierà eventualmente la propria strada verso la salvezza. Tutto questo si ricollega alla centralità della persona umana. La persona e la sua dignità sono il fulcro della storia. Senza tutto questo non c'è Europa. Senza tutto questo si rinnegherebbe la stessa identità europea. Certo, anche l'Europa ha conosciuto l'intolleranza religiosa. È stato il volto peggiore del nostro continente. Anche noi siamo stati capaci di guerre religiose. Abbiamo praticato la discriminazione religiosa perché, anziché un rapporto diretto con la divinità per la salvezza o per il bene dell'uomo, diventava la religione *instrumentum regni*, oggetto di una arrogante supremazia di un uomo su un altro uomo. Anziché momento di elevazione e trionfo della spiritualità, diventa oggetto di dominio e di possesso ed è ciò che purtroppo sta ancora avvenendo oggi. I dati che sono stati citati sono veramente impressionanti. Duecento milioni sono i cristiani che si trovano in una condizione di sostanziale persecuzione. Vi sono Paesi che rinnegano del tutto la possibilità di praticare liberamente i culti, la religione che non siano quelli imposti da un certo ordinamento. la Libia dove il Governo limita fortemente la pratica religiosa, la libertà di culto e l'adesione alla fede cristiana, o l'Arabia Saudita dove persino il possesso della Bibbia è considerato un crimine, o, ancora, la Cina dove i cattolici fedeli al Papa sono considerati agenti di una potenza straniera. tutto questo non è qualcosa che è sempre esistito nei rapporti con un certo mondo diverso da quello europeo, in particolare quello quello musulmano. Infatti, nel corso dei secoli, in Libano, in Spagna o nei Balcani, musulmani e cristiani hanno convissuto insieme, costruendo delle splendide civiltà. Ricordo un dato

se nel 1948 in una città del Medio Oriente l'85 per cento della popolazione era cristiana vuol dire che ci sono state stati anche momenti di convivenza pacifica. non posso non ricordare l'evoluzione che ha caratterizzato altri Paesi. Si pensi ad esempio, al Libano, al dramma recente, di questi ultimi decenni, di 6 milioni di cristiani profughi dispersi nel mondo. E ancora alla Siria. Le comunità cristiane che all'inizio del '900 rappresentavano più di un quarto della popolazione ora sono calate al 7 in questo contesto il germe del fanatismo, dell'integralismo e dell'estremismo sia non soltanto il nemico del Cristianesimo, ma innanzitutto il nemico di quei popoli in cui viene praticato.

all'Europa è importante perché i Paesi appartenenti alla Comunità europea non lascino soli i Governi che lottano contro il fanatismo religioso e, d'altro canto, non appoggino quei Governi che alimentano le persecuzioni, che finanziano i movimenti o i Paesi che legittimano le discriminazioni e le persecuzioni.

Non può lasciare indifferenti il silenzio, a parte qualche isolata eccezione, dell'Unione europea. È ignavia o ignoranza? Quando rinneghiamo il meglio delle nostre radici, della nostra storia, è difficile trovare la consapevolezza di ciò che dobbiamo fare. Allora vanno benissimo gli osservatori sulla libertà religiosa, ma da soli servono a poco.

diciamo che questa Europa, ad iniziare da questa Italia, deve ritrovare l'orgoglio di una grande storia, di una grande testimonianza per contribuire nella pace e nella collaborazione tra i popoli a ridare un futuro un futuro di tolleranza, di civiltà e di progresso alle Nazioni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, intervengo a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, per rappresentare all'Aula, al Paese e a tutti coloro che ci ascoltano il nostro fermo intendimento di condanna assoluta di quanto sta accadendo, da ormai troppo tempo, nei lembi più svariati del pianeta, oggi accomunati da questo forte risentimento anticristiano. Il Senato della Repubblica, in questa legislatura, ha già dovuto occuparsi del problema della persecuzione dei credenti. Già il 26 ottobre 2008 e il 9 dicembre 2009, questo ramo del Parlamento ha voluto impegnare il Governo ad adoperarsi per garantire i diritti fondamentali della persona e le libertà religiose, ponendo fine alle violenze, alimentate dal fondamentalismo etnico religioso, con particolare riguardo alle persecuzioni delle comunità cristiane nel mondo. L'Italia dei Valori, nella mozione che ha presentato e, poi confluita in un documento unitario, ha scelto di sottolineare la gravità delle più cruente violazioni della libertà di culto, di qualsivoglia credo religioso, occorse in questi ultimi anni. Purtroppo la storia, da millenni ormai, narra di violenze, soprusi, morti, guerre o addirittura conflitti mondiali, in nome della persecuzione di comunità religiose, celando dietro questo vessillo più effimeri e fugaci interessi contingenti e terreni. Desidero utilizzare il tempo a mia disposizione per rappresentare la forte preoccupazione circa l'ormai evidente strategia di persecuzione delle comunità cristiane nel mondo. Questa modalità di infierire con il terrore su inermi credenti - rei soltanto del fatto di recarsi in un luogo di culto, come accaduto recentemente ad Alessandria d'Egitto, ma comunque troppo spesso nei Paesi mediorientali oltre ad esser drammaticamente atroce per le modalità con le quali porta la morte, è preoccupante per l'evidente disegno ideologico e di interesse che soggiace alle atrocità medesime. Così come descritto nel testo della mozione, i cristiani oggi - come i tibetani, gli ebrei e decine di altre comunità di credenti prima - rischiano quotidianamente la vita a causa del loro credo religioso e, quando la vita gli è fatta salva, è comunque gravissima la situazione di violenza e discriminazione alla quale sono costretti.

Ma non solo in questi Paesi! Le violenze e i soprusi contro i cristiani, e non solo contro di loro, accadono purtroppo quotidianamente nella quasi totalità degli Stati del globo. L'incremento degli episodi di violenza ed intolleranza a sfondo etnico e religioso coinvolgono infatti anche le società economicamente più avanzate, seppur continui a trovare l'apice nei Paesi nei quali le tensioni politiche e sociali impregnate di fondamentalismo ideologico, qualunque esso sia - sono più forti, come nel caso dei Paesi mediorientali più tristemente noti. Le comunità cristiane di fatto vivono ed operano ormai in una condizione di isolamento e di estraneità rispetto alle dinamiche sociali, politiche e culturali dei Paesi in cui insistono. È un attacco pesante, che ha radici forti e non risparmia nessuno. Le comunità cristiane locali danno fastidio perché con la loro stessa esistenza diffondono una religione, una cultura e un sistema di vita fondati sul valore assoluto della persona umana, quindi sulla libertà, l'uguaglianza di tutti di fronte allo Stato, la donna con gli stessi diritti dell'uomo, la democrazia, la giustizia sociale. Alla politica, cari colleghi senatori

capace di contrastare con efficacia i soprusi perpetrati in ogni angolo del mondo, a danno di uomini e donne di ogni razza o etnia, a causa della professione del loro credo religioso, promuovendo presso gli organismi internazionali e sovranazionali efficaci azioni diplomatiche, esigendo un fattivo ed efficace impegno dell'Unione europea affinché assuma una posizione forte e definita. Credo tuttavia - e questo non sia sufficiente indicare gli accadimenti di questi ultimi tempi e chiedere al Parlamento e al Governo italiano di farsi carico della condanna e delle conseguenti e forti iniziative politiche per risolvere questo dramma. Occorre in questa sede io credo ampliare la riflessione facendoci carico di un diverso, nuovo e autentico impegno nell'attuazione dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, laddove si dice, che «ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione». E allora diventano necessarie alcune condizioni di fondo: democrazia, pace, giustizia, libertà, valori da testimoniare che devono tornare ad essere testimoniati con i comportamenti nella quotidianità, favorendo le aspirazione dei popoli (non con i decreti tampone, cari colleghi), ma con una vera politica di rispetto e non di rapina. Occorre interrogarci sulle ragioni del dialogo e del consenso con i diversi Stati; individuare nella tolleranza un valore condiviso, testimoniato e vissuto in atti concreti. È necessario - io credo - favorire l'abbattimento di quegli steccati che dividono, che sono spesso il frutto della paura dell'altro, del rischio cioè di nuove povertà che inducono ad un nazionalismo oscuro e incapace totalmente di dialogo. Occorre - cari colleghi, passatemi questa mia riflessione - il coraggio di «farsi prossimo», magari emulando un poco quei viandanti di Emmaus che smarriti e attoniti cercavano una risposta. Certo, sono ragioni difficili quelle che noi poniamo, che richiedono fatica, ma non credo vi siano altri percorsi da ricercare per costruire fondamenta solide per una autentica e duratura convivenza umana, recuperando poco a poco le ragioni della credibilità e del rispetto delle idee diverse. Occorre cioè promuovere una ferma condanna dei nuovi egoismi frutto di un modello di sviluppo che porta con sé purtroppo un forte limite ad una legittima speranza per il futuro dei popoli. Onorevoli senatori, io credo che siamo tutti un poco mendicanti di infinito e io credo che il poter esprimere le proprie convinzioni religiose, confrontarle, ascoltarle, viverle, manifestarle sia davvero il modo autentico per celebrare lo stesso concetto di libertà.

a tutti gli stranieri presenti sul territorio italiano che lo abbiano richiesto in quanto vittime, o potenziali vittime, di persecuzioni di carattere religioso nei Paesi d'origine. Signor Presidente, la pacificazione dei popoli passa necessariamente attraverso un percorso che ponga al centro il rapporto tra libertà di religione e tolleranza. La nostra cultura, la cultura cristiana, si fonda sul rispetto del prossimo e delle minoranze in particolare, che vanno tutelate e rispettate. Nel mondo i cristiani non ricevono lo stesso trattamento. Tre quarti delle vittime per motivi religiosi sono cristiani. Di certo, non è facile superare la naturale reazione di indignazione e di rabbia di fronte a questi massacri: quello che ha colpito i cristiani copti in Egitto durante un momento di preghiera è uno dei tanti episodi che hanno lasciato una lunga scia di sangue in diversi Paesi come il Sudan, il Pakistan, il Maghreb e la Nigeria, dove soltanto ieri un attacco ad un villaggio avrebbe causato almeno 13 morti, che si vanno ad aggiungere alle migliaia di vittime degli sconti interreligiosi nell'ultimo decennio. Tutto ciò causa dolore e rabbia, dolore e rabbia, che si provano nel vedere pacifiche comunità oggetto di sterminio. Tuttavia, noi dobbiamo rispondere alla violenza con l'impegno per la pace un impegno da portare avanti con la consapevolezza che la democrazia, per esprimersi pienamente, ha bisogno della libertà religiosa, libertà religiosa che è stata una grande conquista di civiltà delle democrazie di civiltà delle democrazie e va tutelata, difesa e promossa in alternativa ad ogni forma di integralismo e fondamentalismo religioso. Lì dove non esiste libertà religiosa, o in cui essa non è sufficientemente tutelata, si creano indirettamente i presupposti per il diffondersi di forme di estremismo. ciò vale soprattutto per quei Paesi in cui identità nazionale e identità religiosa coincidono, come accade nel mondo islamico, dove alcune forme di integralismo mirano ad affermare che chi non è musulmano non può essere neanche cittadino. Per questo bisogna sfruttare al meglio le relazioni che l'Italia ha in Medio Oriente, affinché fatti come quelli di Alessandria non si verifichino più. Allo stesso tempo è sempre più urgente che l'Italia si faccia promotrice di iniziative presso l'Unione europea e la comunità internazionale perché si agisca concretamente per fermare gli episodi di violenza contro i cristiani nel mondo. Almeno 200 milioni sono i cristiani perseguitati secondo la ACS (Aiuto alla Chiesa che soffre), vale a dire circa quattro volte la popolazione italiana. Onorevoli colleghi, se anche qui in Senato, come alla Camera, abbiamo ritenuto opportuno unificare i testi delle mozioni è perché tutti noi avvertiamo l'urgenza di scuotere le organizzazioni internazionali - *in primis* l'ONU dal torpore e dall'apatia con cui sembrano assistere al massacro dei cristiani, e chiediamo loro un intervento forte e deciso in loro difesa. Il fatto che oggi molte realtà cristiane siano costrette a vivere nel terrore e nel pericolo è un fatto inaccettabile,

della piena reciprocità, cioè offrire rispetto ma anche esigerlo. Come ha detto Papa Ratzinger: «Le grandi religioni hanno contribuito allo sviluppo della civiltà. La sincera ricerca di Dio promuove la dignità umana». Ma siamo

Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghi, purtroppo non è la prima volta che in questa legislatura prendo la parola cercando di attirare l'attenzione dell'Assemblea del Senato su di una problematica che mi ha sempre mortificato come cristiano, come cattolico, come laico e come membro di questa Assemblea. Mi riferisco alle violenze continue perpetrate nel mondo nei confronti dei cristiani che sentimentalmente ormai entrano a far parte della cronaca, ma che la maggiore parte della stampa non sottolinea con la dovuta enfasi. C'è voluto il forte grido di dolore del Santo Padre per riaccendere i riflettori su di una problematica incresciosa facendo capire che la misura ormai è colma. Noto con soddisfazione che molti hanno aperto gli occhi su questa situazione incresciosa, ma non vorrei che questo nostro tempo e queste nostre parole rimangano tracce d'inchiostro sui papiri del Senato senza arrivare a nessuna conclusione concreta, come purtroppo ormai mi sono abituato a riscontrare in molte situazioni nella pur nostra nobile Assemblea. Mi rendo conto che non è e non può essere solo un problema nostro, inteso come problema Paese, ma è giusto per questo che dobbiamo essere dei promotori capaci di sensibilizzare a tutti i livelli istituzionali sul problema della persecuzione dei cristiani, prima, e della libertà religiosa, poi. Sono pienamente convinto però che questa scia di attentati che da troppo tempo perseguitano le varie comunità cristiane non sia un insieme di atti isolati, ma risponda a una strategia frutto di una sola regia mondiale, con obiettivi ben precisi, che trovano poi il loro alimento primario nella perdita di valori che le società, non solo occidentali, continuano a consumare.

usiamo il termine «pace» per sciacquarci la bocca, ma non abbiamo mai fatto cose veramente all'altezza di questo grande valore che dovrebbe essere un obiettivo primario della nostra società e degli uomini tutti; e pensare che il Cristianesimo è la religione per eccellenza dell'amore, ricevendo come risposta il massacro continuo dei suoi componenti e rappresentanti. La pace passa attraverso il diritto di libertà religiosa per tutti gli uomini. Questo diritto lo si può definire universale e riguarda la parte più nobile di una creatura umana, cioè il potersi relazionare con il suo Dio. Se volgiamo il nostro sguardo ai vari continenti non ne troviamo uno che si possa vantare di onorare il diritto alla libertà religiosa. Molto spesso sono gli stessi Governi che inibiscono le pratiche e le espressioni. emblematica la situazione cinese, dove piccole aperture di relazioni tra il Governo comunista cinese e Roma, tempo fa, avevano lasciato credere ad una proficua collaborazione, dando speranza a quei cristiani obbligati ancora adesso a vivere nelle catacombe. Del resto, il passo avvenuto tra novembre e dicembre non fa ben sperare, tanto che si è arrivati a nomine di vescovi senza consultarsi con Roma, rompendo quel rapporto apostolico obbligato per la Chiesa cristiano-cattolica. Se dalla Cina passiamo all'Africa, le note diventano sempre più dolente. Nigeria: possiamo dire che in questa Nazione gli scontri interreligiosi da sempre in atto, e che hanno provocato migliaia di morti, si stanno intensificando. Solo ultimamente gli scontri tra cristiani e musulmani fanno contare più di 1.500 vittime. Di certo il Governo nigeriano ha le sue responsabilità. Pakistan: con un Governo debole come quello che si ritrova, sicuramente gli scontri interregionali fanno da scena e da paravento al terrorismo. Iraq: ancora vive nella mia mente le immagini di quel 31 ottobre 2010 quando un comando di Al Qaeda ha preso d'assalto la cattedrale sirocattolica di Baghdad; a fine giornata si contavano più di 50 morti, compresi donne e bambini. Ma non è finita così: gli attacchi si ripetono, si consumano fin dentro le case dove abitano i cristiani. Ma cosa possiamo dire dell'azione che ha portato Alessandria d'Egitto alla ribalta delle cronache con i tragici fatti del Capodanno? Da subito a me era parsa come una sfida diretta alle parole pronunciate da Benedetto XVI nella Giornata della pace, che il mondo cristiano celebra proprio nella giornata del primo dell'anno. Non dimentichiamo: 29 sono state le vittime ed un centinaio i feriti. I fedeli feriti. I fedeli con spirito amorevole erano raccolti all'interno della loro chiesa e un *kamikaze* accecato dall'odio vi si è fatto esplodere.

di essere stato l'artefice della nostra civiltà, fondata sulla verità e l'amore; ci ha fornito una risorsa stupenda e impareggiabile che ci ha premesso il conseguimento di molti beni, tra cui la dignità della persona umana. Pertanto, l'umanesimo primo e più autentico dell'Europa è quello cristiano. Non dobbiamo dimenticare che le radici cristiane hanno condotto l'Europa alla percezione della verità e al profondo rispetto dell'uomo. All'origine della Comunità europea e del Trattato di Roma del 1957 si trova iscritto il concetto fondamentale di comunità nata dalla tradizione cristiana. Più chiaramente, l'Europa dei diritti e dei doveri deve la sua esistenza al Cristianesimo, vedendo la luce il giorno stesso in cui l'uomo, da Tertulliano in poi, ha posto in rilievo la dignità della persona umana nella ricerca della verità, della giustizia, della libertà e più tardi nel rispetto dei diritti di ogni uomo. Come dicevo in precedenza, il grande bene che il Cristianesimo può elargire alle società nuoce a quelle forze del materialismo unite sotto il vessillo della Babilonia che marciano compatte per distruggere i nuclei di spiritualità cristiana vivente. Le colpe non possono che essere nostre. Dobbiamo dichiarare le nostre radici cristiane con decisione partendo dalla Carta costituzionale europea: tutti noi dovremmo recuperare quei valori che il secolarismo ci sta facendo perdere. Voglio fare una riflessione sugli incidenti occorsi a Roma durante le manifestazioni universitarie. I magistrati hanno liberato i ragazzi il giorno dopo il fermo perché erano incensurati. Ma dov'erano le famiglie di questi ragazzi? A casa mia, alla mia età, non avrei potuto tornare dai miei genitori dopo aver compiuto tali misfatti. È il secolarismo della nostra società che porta a queste distruzioni. Non dobbiamo aver vergogna di dichiararci cristiani e di sottolineare tutti i valori

la comunità internazionale non può essere cieca ancora una volta. L'evento non può essere dissociato dagli attacchi massicci contro i cristiani di tutte le confessioni nei Paesi a maggioranza religiosa diversa, per lo più islamica ma anche induista. La lista nera delle azioni anticristiane va dal Sudan alla Nigeria, dal Medio Oriente alla penisola arabica, dal Pakistan all'India fino alla storia drammatica di Timor Est, in Indonesia. I cristiani copti in Egitto, come tutte le altre importanti comunità cristiane in Medio Oriente, sono una comunità di antichissima tradizione. La loro esistenza risale alla prima età del Cristianesimo, molti secoli prima della nascita dell'Islam, e gli imperi e le autorità islamiche che si sono succeduti nel territorio hanno sempre accettato la loro presenza. Mette conto sottolineare la particolare tolleranza mostrata da uno dei maggiori imperi islamici della storia, quello dei turchi ottomani, rispetto alle minoranze cristiane (ed ebraiche) non solo dell'Egitto, ma anche del Medio Oriente, dell'Anatolia e dei Balcani. Il sistema di convivenza e di regole garantito per secoli ha subito una grave crisi con il crollo dell'Impero ottomano agli inizi del Novecento e con i sommovimenti concomitanti alla Prima e alla Seconda guerra mondiale. In seguito, i contradditori fenomeni del post-colonialismo non hanno fatto altro che aggravare le tendenze all'intolleranza e al rigetto, e in molti Paesi la componente cristiana si è drasticamente ridotta. Oggi i propugnatori dell'integralismo islamico mirano a far precipitare la situazione e ad introdurre una rottura radicale rispetto alla storia e alle stesse prospettive future. L'obiettivo degli integralisti è la creazione di una società totalmente omogenea, ma di questo processo di islamizzazione integrale ad essere vittime non sono soltanto cristiani, ebrei o induisti; sono anche, e spesso soprattutto, gli stessi islamici: islamici considerati "eretici" o "eterodossi"; islamici che cercano una sintesi creativa fra la loro confessione e il pensiero occidentale; islamici che cercano una strada originale verso il pensiero laico. Nella stessa società e cultura egiziana oggi si sottolinea che l'attentato di pochi giorni or sono è contemporaneamente un attacco ai cristiani, agli islamici e soprattutto all'Egitto, che diventa un paradigma di ciò che sta accadendo in questi anni della globalizzazione nell'area islamica. motivo? Perché la convivenza, anche in forme conflittuali, di comunità culturalmente e religiosamente distinte appartiene da sempre alla storia dell'Egitto e alla sua stessa identità. Dietro all'attacco materiale, l'attacco simbolico è altrettanto grave: è l'attacco alla convivenza delle diversità, siano esse religiose, etniche, linguistiche, culturali. Dinanzi a chi asserisce l'inevitabilità dello scontro di civiltà, e si adopera per precipitarlo, dobbiamo asserire vigorosamente che quello che attualmente ha luogo è uno scontro entro ciascuna civiltà, che taglia trasversalmente ciascuna confessione, ciascuna cultura, ciascuna Nazione; è lo scontro che concerne opposte visioni della convivenza e dell'interazione fra confessioni, fra culture, fra Nazioni: fra coloro che ritengono la convivenza e l'interazione essenziali per il presente e il futuro di tutte le comunità e coloro che le vorrebbero senz'altro eliminare. Non c'è dubbio che la violenza fondamentalista rappresenti la risposta più regressiva e distruttiva alle sfide della globalizzazione, quella della chiusura in un'identità contrapposta alle altre identità. La storia, al contrario, ci insegna che le identità più capaci di diventare fonte di civiltà sono quelle che rinunciano all'imposizione violenta e ideologica, traendo la loro sostanza dal confronto con le altre identità e civiltà. Il mondo globalizzato richiede più che mai da parte nostra, in particolare italiani ed europei, una piena accettazione e un rafforzamento di questa logica di apertura, che non significa rinuncia alla propria identità e alla propria storia, ma - nel caso dell'Europa - la sua autentica realizzazione. Questa del resto è la conclusione matura a cui è giunto il cristianesimo, dopo una storia lunga e difficile, che in molti casi lo ha visto contrapposto ad altre religioni e culture. Ed è anche la lezione che l'Italia e l'Europa hanno saputo ricavare dagli errori del loro drammatico passato. In Europa, come sappiamo, la libertà religiosa non è una realtà originaria. È stata una lenta conquista nell'ambito di un lungo processo storico, dopo che le guerre di religione intracristiane avevano mostrato i loro esiti distruttivi ed involutivi. E la presa di coscienza dell'essenzialità della libertà religiosa è stato un grande progresso, un punto di non ritorno per il pensiero laico e per le grandi confessioni cristiane,

fra tante fatiche e tante ferite. Questa è effettivamente un'eredità globale dell'Europa, alla quale si appellano tanti individui e tante collettività anche esterni alla cultura e ai modi di vita occidentali (pensiamo solo alla lunga lotta per i diritti condotta con vigore da tante donne nel mondo islamico), quale precondizione di una condizione globale che consenta a tutti, soprattutto nell'età della globalizzazione, di convivere e di fiorire insieme. Per tale ragione, a nome del Gruppo del Partito Democratico, esprimo la soddisfazione di poter sostenere un documento condiviso da tutti i Gruppi parlamentari. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, credo sia stata opportuna la scelta di discutere oggi nel Parlamento italiano della cristianofobia e degli eventi che recentemente hanno colpito l'opinione pubblica internazionale e, in particolare, l'Italia.

Noi apprezziamo gli sforzi in atto del Governo egiziano affinché siano assicurati alla giustizia gli autori di questo efferato episodio e confermiamo il sostegno e l'amicizia a quel Governo impegnato in una difficile opera di contrasto al terrorismo che colpisce

affinché, come ha evidenziato nei giorni scorsi il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Bagnasco, «la comunità internazionale faccia sentire una voce forte ed una parola chiara perché il diritto alla libertà religiosa sia osservato ovunque senza eccezioni». una vasta dottrina che appartiene al diritto pubblico ed al diritto internazionale ha affermato che la libertà religiosa costituisce una delle basi fondanti dei diritti della persona umana. Ciò spiega perché la libertà di religione sia inserita in maniera chiara nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Il diritto codifica quanto è stato già riconosciuto dalla filosofia e dal libero pensiero: non c'è libertà in senso lato senza libertà religiosa. La libertà di religione, in altre parole, è parte integrante dell'essere uomini e donne liberi. Nell'articolo 8 della nostra Costituzione si afferma: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti». Questa consacrazione chiara e decisa al punto di trovare forza nella suprema legge indica che per noi la libertà religiosa è un valore garantito a tutti, ovviamente anche a chi appartiene a confessioni religiose diverse da quella cui è legata la nostra tradizione di popolo e di nazione, cioè la Chiesa cattolica. Vale la pena ricordare che la formulazione dell'articolo 8 rappresenta un passo in avanti rispetto a quella del vecchio statuto che parlava semplicemente di culti tollerati. La libertà religiosa intesa come possibilità concreta di esercitare la propria fede è un dato irrinunciabile della persona e, se la si nega, si porta un'offesa alla dignità umana. Il fatto decisivo che noi riconosciamo la libertà religiosa come valore costituzionale significa che per coerenza dobbiamo essere pronti anche ad un impegno forte e severo affinché la libertà religiosa sia garantita ovunque nel mondo. L'Occidente ha elaborato una teoria della sacralità dell'uomo che pone al centro dell'idea di democrazia la sacralità dell'individuo portatore di diritti e di doveri; lo sviluppo di questa idea non sarebbe stata possibile senza l'apporto del Cristianesimo, che ha influenzato positivamente il germoglio della libertà nelle nostre società. In passato l'Italia si è impegnata con la sua politica internazionale contro le dittature che in ogni parte del mondo hanno oppresso anche il mondo cattolico e tante vicende internazionali richiamano la passione civile con cui l'Italia si è battuta su questi fronti. Per gli stessi motivi di allora, oggi la nostra politica estera deve lavorare per il rispetto concreto e attivo della libertà di religione in ogni parte del pianeta,

con il diritto della Convenzione, proprio perché minaccia la libertà religiosa. *(Applausi della senatrice Bonfrisco).* L'Italia deve agire affinché l'Europa tenga fede ai suoi principi, a quei principi morali che si è liberamente scelta e che sono ampiamente condivisi. Parlammo di questi argomenti, qui in Senato, quando il 30 ottobre del 2008 sottoponemmo all'Assemblea una mozione relativa all' orrenda strage che, nello Stato di Orissa, in India, aveva colpito dei cristiani. Tutto il Senato condivise quella mozione e prese una posizione decisa per spingere il nostro Governo alle adeguate iniziative internazionali. Voglio ricordare soprattutto la sottovalutazione, fanno solo le organizzazioni internazionali, ma che spesso tutti noi facciamo nei confronti delle persecuzioni dei cristiani. La comunità internazionale è insorta in tanti casi, anche famosi, di lapidazioni minacciate o di crimini orrendi, che vanno ovviamente contestati e contrastati: è dunque stata giusta la nostra mobilitazione. I fenomeni di cristianofobia non hanno però suscitato la stessa reazione e la stessa emozione, perché c'è stata troppa assuefazione o troppa rassegnazione.

in questa iniziativa concreta. L'ordine del giorno dà infatti indicazioni precise al Governo per prendere iniziative nelle sedi internazionali affinché l'Europa - e non solo l'Europa - agisca perché la libertà religiosa venga garantita in ogni parte del mondo.

certamente una dimensione di arricchimento della persona. Il Santo Padre ha ricordato che in tante parti del mondo «la vita delle comunità religiose è resa difficile e talvolta precaria perché l'ordinamento giuridico o sociale si ispira a sistemi filosofici o politici che postulano uno stretto controllo, per non dire un monopolio, dello Stato sulla società»: è stato ricordato il caso della Cina o di altre parti del mondo in cui la libertà religiosa viene conculcata. «Il peso particolare di una determinata religione in una nazione non dovrebbe mai implicare» ha detto Benedetto XVI «che i cittadini appartenenti ad un'altra confessione siano discriminati nella vita sociale o, peggio ancora, che sia tollerata la violenza contro di essi». Il Pontefice ha ricordato l'importanza del dialogo interreligioso, che possa favorire «un impegno comune a riconoscere e promuovere la libertà religiosa di ogni persona e di ogni comunità». Sono state infatti annunciate, per i prossimi mesi, nuove iniziative in questa direzione. Riteniamo dunque che non ci si debba limitare a un atto di circostanza

proprio, ha ricordato come questa discussione avvenga a dieci anni dal 2001, anno caratterizzato da drammatici, devastanti, tristemente storici eventi di intolleranza. Vogliamo operare per un mondo in cui

iniziative concrete. Siamo certi che, anche dopo il dibattito odierno, l'unità del Parlamento su questa altissima sfida di libertà, di civiltà,

richiamare l'attenzione dei mezzi di comunicazione, ma che, accanto alle iniziative dei liberi Parlamenti, dei Governi e delle organizzazioni internazionali, tutti debbano fare propria questa grande battaglia di civiltà.

noi senatori Radicali ci asterremo nel voto su questo ordine del giorno, non tanto e non solo perché non condividiamo alcuni degli elementi e dei meccanismi operativi che vengono chiesti, ma in sostanza e soprattutto perché non condividiamo l'analisi che viene fatta sottintende, in particolare per quanto riguarda l'Egitto o l'Iraq. Non nego, al contrario, che siano in corso vere e proprie campagne contro la libertà religiosa, in particolare contro i cristiani, e mi dispiace molto, ad esempio, che nell'elenco contenuto nella mozione non siano indicati i Montagnard, che sono la comunità vietnamita più

Quello che sta avvenendo in Egitto è in realtà uno scontro interno alle varie famiglie dell'Islam - quella più militante, quella più dialogante e quella più istituzionale - ed è un problema altamente politico: sono gruppi che fanno politica, di cui i copti sono drammaticamente vittime, ma quasi casuali, perché quello che si registra è invece la volontà politica

dove in realtà il problema è quello di una transizione di regimi autocratici antichi ed obsoleti senza adeguate garanzie. Da laica

Ma quello che contesto è l'analisi sottintesa a questo ordine del giorno. È vero che in Iraq - ad esempio - c'è stato un esodo di cristiani, ma come risultato di un clima di paura e di instabilità dovuto ad uno scontro senza quartiere tra sciiti e sunniti.

Sono in corso campagne cristianofobiche o islamofobiche. In altre regioni sono in corso, ed è tuttora in corso, uno scontro senza quartiere, di potere, tra le varie famiglie islamiche, nel quale i copti sono vittime di paura e di destabilizzazione, con conseguenze drammatiche; ma l'obiettivo è un altro. L'obiettivo è esattamente la destabilizzazione delle parti politiche, magari autarchiche, oligarghiche o anche autoritarie, ma certamente non di stampo combattente. Quindi, diversa attenzione dovremmo prestare anche in promozione della libertà religiosa in alcune grandi zone del mondo, rispetto ad altre dove la motivazione di questi eccidi è completamente diversa. *(Applausi delle

Signor Presidente, intervengo per ricordare all'Assemblea un questione e per chiedere che venga messa in discussione una mia proposta di legge relativa al Patto di stabilità,

che purtroppo ha un meccanismo assolutamente schizofrenico; pensate che questa amministrazione ha avuto un avanzo di gestione di 314.000 euro nel 2004, di 271.000 euro nel 2005, di 1.264.000 euro nel 2006, di 165.000 euro nel 2007, di 308.000 euro nel 2008 e di 101.000 euro nel 2009. il meccanismo perverso del Patto di stabilità prevede che questo Comune, nell'anno in corso, dovrebbe accantonare 1.400.000 euro rispetto all'avanzo che ha già prodotto negli anni precedenti.

a qualcuno in quest'Aula dia fastidio che si ricordi che la 'ndrangheta purtroppo c'è anche in Lombardia e nella provincia di Milano, ma è così; infatti molti sindaci leghisti stanno rimarcando questo fatto chiedendo al presidente Formigoni di rimuovere la nomina. Anche se non è provato, anche se è solo un sospetto, perché tra le nomine discrezionali di carattere fiduciario del Presidente - come ama sempre ripetere lui - ci debba essere una persona che sta suscitando questi dubbi, queste perplessità e questo scandalo

*(IdV)*. Signor Presidente, desidero informare i colleghi che ieri è stata pubblicata un'importante sentenza la n.7674/ 2010 emessa dalla prima sezione del tribunale di Torino (dottoressa Stefania Tassone), che ha condannato una banca, Intesa Sanpaolo, a risarcire 474.000 euro, oltre le spese legali, a una famiglia indotta ad investire tutto il proprio risparmio in titoli tossici della Lehman Brothers pubblicizzati con il bollino della massima affidabilità sul sito della ABI PattiChiari che, al contrario, riteneva rischiosi i titoli di Stato come i BTP. È una sentenza importante, signor Presidente, colleghi, che oltre ad accogliere le tesi dell'avvocato Cecilia Ruggeri, delegata ADUSBEF di Torino, censura pesantemente i consigli degli acquisti dell'ABI che, mediante il consorzio Patti Chiari, suggeriva di acquistare titoli tossici alle famiglie, bollinandoli con la tripla A anche all'indomani del 14 settembre 2008, data del *crack* della banca dei fratelli Lehman. È molto importante diffondere il contenuto di questa sentenza, pubblicato sul sito "www.adusbef.it", che menziona alcune perizie acquisite dai tribunali secondo le quali le banche, già dal gennaio 2008, quasi nove mesi prima del *crack* della Lehman, erano perfettamente al corrente dell'imminente fallimento,

che dopo avere criticato gli eccessi dei banchieri ed i *bonus* esagerati, ha capitolato facendo un'ingloriosa retromarcia e lasciando che i "*bankster*" di Downing Street deliberassero 8,5 miliardi di euro di *stock option,* dopo che la Royal Bank all'83 per cento di proprietà dello Stato inglese, ha ricevuto 45 miliardi di euro per evitare il fallimento.

misure di contrasto all'avidità dei banchieri, anche di casa nostra, che rappresentano la principale causa delle macerie, dei crack e dei fallimenti, con 30 milioni di posti di lavoro distrutti dal 7 luglio 2007, per loro esclusiva avidità e smisurato egoismo. Di tali questioni, signor Presidente, ritornerò ancora a parlare perché la gente che ha rischiato il risparmio sudato di una vita per i cattivi consigli delle banche che hanno indotto ad ad investire nei titoli Lehman o in altri titoli tossici possa riscattarsi anche con il nostro aiuto. *(Applausi dai

L'interrogazione afferisce al pericolo che nelle acque circostanti l'isola di Pantelleria e in altre zone del Mediterraneo prospicienti le nostre coste possano essere effettuate trivellazioni petrolifere su concessioni rilasciate dai Paesi rivieraschi, in con l'acquiescenza del Governo italiano. Siccome la questione è estremamente sensibile ed è avvertita con grande preoccupazione dalle popolazioni di quelle isole e dell'intera Sicilia,